del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria"

sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 giovedì 8 febbraio, alle ore 12,30, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

La relatrice, senatrice Bongiorno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Presidente, svolgerò questa relazione in forma sintetica e poi depositerò agli atti una relazione più completa. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, che è stato approvato con una serie di modifiche dalla Commissione giustizia in sede referente. Il disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, quindi si tratta anche di una serie di norme eterogenee, che cercherò brevemente di illustrare. Gli articoli sono nove. La linea di intervento è riconducibile a tre obiettivi: da un lato si fanno, come dicevo, modifiche al codice penale, in materia di giustizia penale, ordinamentali e di interpretazione autentica. Comincerei con le modifiche al codice penale: l'articolo 1 interviene in materia di delitti contro la pubblica amministrazione; viene abrogato il reato di abuso d'ufficio e viene riscritta la disciplina del traffico di influenze illecite. Su questo nuovo reato facciamo qualche piccola precisazione. Viene previsto che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere utilizzate e non soltanto vantate,

l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, dev'essere economica. E ancora, la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altre utilità economiche sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio o di uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita. Viene aumentato il trattamento sanzionatorio e il minimo edittale passa da un anno a un anno e sei mesi. Ricordo, proprio con riguardo alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, che la Commissione ha già approvato un ordine del giorno con il quale

penale, relativo alle garanzie di libertà del difensore. Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, viene, da un lato, esteso il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato dall'altro, viene introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate. Ci sono ulteriori modifiche che riguardano la disciplina delle intercettazioni. Viene ampliato infatti il divieto di pubblicazione del contenuto delle operazioni captative, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. La riforma interviene anche sulla disciplina delle modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo il divieto di riportare nei verbali espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare i soggetti diversi dalle parti. parti. Corollario dell'intervento sulla disciplina in tema di modalità esecutive delle intercettazioni è una modifica che la Commissione ha apportato all'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di archivio delle intercettazioni. modifica, il procuratore della Repubblica sarà tenuto a impartire, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio, le prescrizioni necessarie a garantire anche la tutela del segreto sui dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. C'è poi un intervento in tema di misure cautelari: per meglio tutelare la *privacy* degli imputati è previsto il divieto per il pm di indicare nella richiesta di misura cautelare con riguardo alle intercettazioni i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo ovviamente che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. Ricordo ancora che sono di indubbio rilievo l'introduzione dell'istituto dell'interrogatorio preventivo del soggetto richiesto dalla misura cautelare, cautelare, precisando che il contraddittorio anticipato è però escluso quando ricorre il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o se si tratti di reati gravi, commessi con l'uso delle armi o altri mezzi di violenza personale. Ricordo ancora la collegialità della decisione quando la misura riguarda una custodia cautelare in carcere o una misura di sicurezza detentiva. Preciso che l'operatività della collegialità è differita di due anni all'esito del reclutamento straordinario di magistrati. Sempre con riguardo alle tematiche processuali, si devono ricordare le modifiche della disciplina dell'informazione di garanzia, che dovrà contenere una descrizione sommaria del fatto; la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato e l'esclusione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti per reati a citazione diretta. Infine, con riguardo al terzo e ultimo profilo di intervento, il disegno di legge reca una norma di interpretazione autentica della legge n. 287 del 1951, per la quale il requisito anagrafico di sessantacinque anni di età, previsto per i giudici popolari delle corti d'assise, si deve intendere riferito al momento della nomina. In conclusione, il disegno di legge oltre a prevedere il citato reclutamento straordinario di magistrati, interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari.

una di queste si ha quando il pubblico ufficiale intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto. Tale abuso si può realizzare in due modalità: con l'emanazione di un atto oppure con un comportamento materiale. Quando l'abuso si consuma con un comportamento materiale, non è possibile rivolgersi al giudice amministrativo, quindi si verifica una lesione del diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione, che stabilisce che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi». Ebbene, i cittadini che subiranno un abuso d'ufficio con comportamenti materiali non avranno più la possibilità di rivolgersi a un giudice. È interessante notare che la casistica delle condanne definitive per abuso d'ufficio, dal 1996 al 2020, ha evidenziato diversi casi di condanna definitiva per abuso commesso con comportamenti materiali. il declassamento di questi comportamenti prevaricatori di condotte che oggi integrano un reato in fatti che hanno rilievo solo sul piano etico-sociale la conseguente disattivazione deterrente della sanzione penale assumono il significato di un riorientamento culturale in senso negativo, perché liberalizza tutti i comportamenti di abuso - che oggi sono penalizzati degradando il livello della pubblica amministrazione. Si configura in questo modo la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che tutela il principio del buon andamento e dell'imparzialità, e dell'articolo 54 della Costituzione. Abbiamo anche un altro profilo. L'abolizione dell'abuso d'ufficio nei casi nei quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una palese violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione, legittimando quindi l'uso dell'azione penale per la tutela di questo bene. La violazione di tale articolo della Costituzione appare tanto più rilevante ove si consideri che la disattivazione della sanzione penale si somma all'assoluta inadeguatezza della legislazione attualmente vigente in materia di conflitto di interesse com'è stato rilevato in varie sedi istituzionali - e all'assoluta mancanza di una legge sulle *lobby*. La sinergia negativa tra la disattivazione della repressione penale dell'abuso d'ufficio per conflitto di interessi e questi altri fattori crea quindi l'*habitat* ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'articolo 97 della Costituzione. Ancora, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di abolire questo reato, che si concreta in una pluralità di condotte, tra le quali anche l'intenzionale strumentalizzazione del potere pubblico per finalità approfittatrici, sopraffattrici e prevaricatrici, contemporaneamente mantenendo invece in vita il reato di omissione di atto d'ufficio, previsto dall'articolo 328

Altro profilo di incostituzionalità: l'abolizione dell'abuso d'ufficio, basata sulla *ratio* di evitare la cosiddetta paura della firma, è assolutamente priva di ogni ragionevolezza, tenuto conto che, come tutti i giuristi sanno, a seguito della riforma del 2020, è stato eliminato ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia sfera dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione ed è rimasta punibile soltanto la violazione di norme imperative e cogenti derivanti dalla legge, che non lasciano alcun margine di discrezionalità. L'abolizione del reato, anche quando vi sia la violazione intenzionale e profittatrice di norme cogenti da cui non residua alcun margine di discrezionalità, configura quindi una violazione palese dell'articolo 3 della Costituzione per l'incongruenza del mezzo (l'abolizione del reato) rispetto al fine. l'abrogazione dell'abuso d'ufficio configura una violazione dell'articolo 117 della Costituzione, avuto riguardo alle gravi ricadute immediate sull'attività della procura europea, organismo indipendente dell'Unione europea operativo dal 2020 e incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Quest'attività della procura europea assume un rilievo particolarmente importante in questa fase storica, nella quale sono in ballo 195 miliardi del PNRR. Ebbene, l'abolizione dell'abuso d'ufficio determina, come effetto immediato, l'archiviazione di tutti i procedimenti penali in atto pendenti presso la procura europea e la disattivazione per il futuro dell'esercizio dell'azione penale da parte della procura europea per tutti i reati d'abuso d'ufficio che determinano una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Questo viola l'articolo 117 della Costituzione, con riferimento all'articolo 83 del testo unico del funzionamento dell'Unione europea. Un'altra norma che presenta profili di incostituzionalità è l'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, di questo disegno di legge, che elimina la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello, nei casi di proscioglimento dell'imputato, quando si proceda per delitti per i quali l'azione penale viene esercitata mediante la citazione diretta a giudizio. Ora, vorrei far rilevare ai senatori che, anche a seguito della riforma Cartabia, l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede la citazione diretta per reati puniti sino a dieci anni di galera: il furto pluriaggravato, la ricettazione (punita sino a otto anni di galera) o le lesioni stradali gravissime (punite sino a sette anni di galera). allora che qui si viene a verificare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione; non si comprende per cui imputati prosciolti per questi reati gravissimi (puniti sino a dieci anni di galera) debbano godere del privilegio di vedere non appellabile la loro sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero, mentre altri invece prosciolti invece prosciolti per reati meno gravi, per i quali è prevista non la citazione diretta, ma l'udienza preliminare, puniti sino a quattro anni e mezzo di galera, come il traffico di influenze ed altri, invece non possano godere dello stesso privilegio accordato a imputati è assolutamente irrazionale anche perché questa norma è palesemente contraria ai principi della Corte costituzionale, che ha già bocciato la legge Pecorella, che aveva precluso al pubblico ministero la possibilità di presentare appello nei casi di proscioglimento per giudizio abbreviato.

dell'ascolto, a parlare di questioni di legittimità costituzionale nella giornata in cui i cancelli del carcere di San Vittore sono stati chiusi alla Costituzione.

di fare quello che sarebbe invece auspicabile, cioè discutere di cosa vuol dire essere cittadini. E questo dopo quel bellissimo viaggio che la Corte costituzionale aveva fatto nei luoghi importanti del nostro Paese, nei luoghi esistenziali e fisici, a partire dalle scuole e dalle carceri. Tuttavia, l'ottimismo della volontà mi spinge comunque a entrare nell'argomento. Vi sono una serie di premesse che vanno fatte, parlando dell'abolizione totale del reato di abuso d'ufficio, rispetto

non renderebbe impossibile l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ovvero l'inizio di un'indagine, perché, a fronte di una denuncia, comunque

Il Partito Democratico ha avuto sempre molta attenzione su questo tema, in particolar modo anche alle preoccupazioni degli amministratori. Da un lato, già nel 2020, com'è arcinoto, era stata ridotta la portata della fattispecie, con una giurisprudenza assolutamente maggioritaria e costante che ne dà riscontro. Naturalmente, ci possono essere ipotesi migliorative. I nostri emendamenti andavano esattamente in questo senso, ma sono stati respinti senza neanche essere stati presi in esame, a conferma di un approccio molto propagandistico ed ideologico, che non ha niente a che vedere con i timori degli amministratori. Infatti, giacciono dalla scorsa legislatura, ripresentati in questa, due proposte di legge a nostra firma sulle altre e ben più preoccupanti responsabilità per gli amministratori, cioè i reati omissivi impropri, il danno erariale e financo la modifica di quella parte della legge Severino sulla sospensione dalla carica con una sentenza non definitiva (ovviamente, dal nostro punto di vista, escludendo reati di stampo mafioso e reati più gravi); quindi numerose le proposte emendative che non sono state prese in esame, come dicevo. Arrivo solo per ultima alla questione dell'Europa, che ovviamente ci richiama a uno dei profili C'è preoccupazione nelle sedi europee e segnaliamo che ovviamente non sono destinate ad avere successo le affermazioni del Ministro della giustizia, per cui basta cambiare un po' l'ordine delle priorità e anche le sedi europee non potranno che convenire: basta cioè cambiare qualche formalismo e anche la valutazione può cambiare. Naturalmente, mi richiamo all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa dev'essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ora, in questo campo come in altri,

secondo, perché ormai le dimensioni internazionali impongono di tenerne conto e di dare un contributo da protagonisti. Invece noi in questo campo, come in altri, stiamo vedendo parallelamente una discussione di natura economica fondamentale; chiamandoci fuori dal «ce lo dice l'Europa» non possiamo che subirne le iniziative e rinunciamo a un ruolo da protagonisti. Veniamo però al punto: il «ce lo dice l'Europa» sta in un fatto fondamentale, cioè che l'abuso del pubblico ufficiale, per per tradizione dello Stato di diritto, non può essere tollerato e non può lasciare il cittadino privato in balia di qualsiasi abuso. Questo - mi permetto di dirlo ancora una volta - rientra nella cultura garantista, autentica e storicamente consolidata di non abbandonare qualsiasi cittadino a qualsivoglia abuso. Seconda questione:

cittadini comunque sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi esercita funzioni pubbliche, quindi in una posizione di supremazia, che non vi sarebbe in alcun modo sottoposto.

che vorremmo fossero ricordate non soltanto quando si parla dell'Europa dalle radici cosiddette cristiane, perché c'è un'Europa liberaldemocratica, che nasce soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, della quale tutti dovremmo sentirci culturalmente partecipi. Avviandomi alle conclusioni, su questo punto specifico i dati del Ministero ci dicono che la stragrande maggioranza delle ipotesi di reato che vengono iscritte e giudicate non riguardano i pubblici amministratori, ma riguardano altri funzionari, a partire addirittura dagli stessi magistrati. Passiamo alle altre ipotesi di illegittimità costituzionale, come quella sul traffico di influenze, laddove si restringe alla sola utilità economica: da questo punto di vista, si priverebbe il controllo su tutti i favori non economici che invece sono assolutamente sottostanti a rapporti del tutto illeciti. c'è la questione dell'appello del pubblico ministero, che è stato affrontato in modo a dir poco grossolano e incurante delle sentenze della Corte costituzionale e finanche finanche dei lavori della cosiddetta Commissione Lattanzi, che in una sua iniziale proposizione teneva conto del quadro costituzionale, temperando e non creando disparità di trattamento. Per non parlare del fatto che, com'è appena stato ricordato, ricordato, non sarebbe più appellabile una serie di reati che vengono sbandierati da parte di questa maggioranza, quando si ricorda che bisogna assolutamente marcire in galera (i reati che ci vengono ricordati più spesso sono i furti aggravati in appartamento, le truffe e quant'altro, che ovviamente rientrerebbero in questa previsione). Questi sono i profili di illegittimità costituzionale che sono assolutamente inequivocabili, ma che ci rimandano anche a un quadro d'insieme che dovrebbe imporre quella ragionevolezza e quell'approccio cauto, ponderato e anche attento alle obiezioni che vengono sollevate quando si parla di ipotesi di reato e di norme di norme di procedura che riguardano la libertà dei cittadini, ma anche il fatto che un processo possa andare a buon fine. È un approccio che vediamo totalmente assente

che, se non sono inutili, sono comunque dannose per il sistema. È un'altra occasione persa per parlare di giustizia e di diritti dei cittadini.

colleghe e colleghi, abbiamo ritenuto di presentare una questione pregiudiziale su questo disegno di legge e chiedervi quindi di fermarne l'approvazione perché crediamo che violi la Costituzione sotto svariati profili. Innanzitutto, la scelta di abrogare l'abuso d'ufficio contrasta con i principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Questo reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale: rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, ovviamente. L'argomento secondo cui a motivare l'intervento legislativo sarebbe il basso numero di condanne dibattimentali non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie colleghi, è la scarsa tassatività della fattispecie, compito del legislatore sarebbe quello di correggerla, non di cancellarla dall'ordinamento. Come segnalato da buona parte degli auditi, tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione più gravi. In secondo luogo, l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, sulla stessa linea della Convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione che, all'articolo 11, impegna gli Stati membri a prevedere come reato Un altro profilo di incostituzionalità riguarda l'evidente violazione dell'articolo 21, che tutela la libertà di stampa. Questa è una vera e propria legge bavaglio, cari colleghi, e, come se non bastasse, gli interventi in materia di intercettazione a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento, di cui all'articolo 2, comma 1, pregiudicano altresì l'esigenza del diritto di difesa dell'indagato, di cui all'articolo 24 della Costituzione, non essendo egli messo in condizione di conoscere le compiute generalità dei soggetti che con lui hanno interloquito e che di lui hanno parlato nelle conversazioni captate. In ultimo, nel prevedere l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità, il disegno di legge si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, perché comporta una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza, sia rispetto all'articolo 27,

n° 26) la Corte segnalò: la lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost. (consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»); il contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; diritti»; la violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di

formulate dalle opposizioni, che si basano sostanzialmente su due rilievi. Il primo rilievo concerne l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. L'opposizione sostiene che in questo caso l'*abrogatio criminis* sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. I motivi che abbiamo sentito poc'anzi esposti sono, a nostro giudizio, del tutto infondati. La Corte costituzionale ha precisato più volte che definire il perimetro normativo dei reati è competenza esclusiva del legislatore, non sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente irragionevole. Nel caso in esame, a chiedere l'abrogazione del reato sono i sindaci di tutti i colori politici, PD compreso, e lo ricorderemo poi anche in discussione generale. Difficile, quindi, è sostenerne la manifesta irragionevolezza. L'*abrogatio criminis* non evita, inoltre, che l'eventuale abuso sia censurabile in sede amministrativa o contabile. Non c'è dunque alcuna violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro, è proprio l'attuale formulazione del reato di abuso, variata più volte nel corso degli anni e sempre in modo insoddisfacente, a porsi in contrasto con i principi di tassatività e legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione. Infatti, come segnalato in tante occasioni, il reato di abuso è un reato a condotta evanescente, in cui il confine tra lecito e illecito è sempre stato nebuloso e generico. È un reato che si è sempre prestato a interpretazioni giurisprudenziali divergenti e non uniformi. L'abolizione del reato, dunque, non è incostituzionale, semmai piuttosto sana un *vulnus* costituzionale. Il testo di legge viene criticato per un secondo motivo: motivo: proponendo per alcuni reati minori la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, si esporrebbe alle stesse censure che portarono alla dichiarazione di incostituzionalità della legge Pecorella. Tale argomentazione può essere confutata sotto diversi profili che andrò a illustrare. La sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, con cui è stata a suo tempo dichiarata con cui è stata a suo tempo dichiarata l'incostituzionalità della legge Pecorella e che oggi le opposizioni citano a sostegno delle loro tesi, appare viziata da molti punti di vista che andremo a esporre. Intanto, come premessa, essa va collocata in un preciso contesto storico, è stato tutt'altro che ininfluente sull'esito finale del giudizio di legittimità costituzionale: era il periodo del furore ideologico contro il Governo Berlusconi; era il periodo del "resistere, resistere, resistere", e ricordiamo tutti le parole del procuratore Borrelli. Ogni iniziativa in materia di giustizia veniva bollata di fronte all'opinione pubblica come legge *ad personam* e, come tale, da cancellare appena possibile. Per noi è evidente che in quel particolare contesto anche la Corte si è lasciata condizionare dal surriscaldato clima politico ed è pervenuta a conclusioni giuridiche che non esitiamo a definire quantomeno opinabili e comunque viziate dal pregiudizio ideologico. Passiamo ora a esaminare la sentenza della Corte nel merito. La sentenza del 2007 si fondava in via principale sul concetto di assoluta parità tra accusa e difesa, previsto dall'articolo 111 della Costituzione. E già qui possiamo cominciare a discutere. Nel processo civile è sempre così: esiste una piena eguaglianza delle armi tra attore e convenuto, ma nel processo penale, invece, vanno fatti opportuni distinguo. La migliore dottrina ci spiega che nel processo penale parità significa non identità, ma equilibrio dei poteri. La parità, evidentemente, attiene alla sola fase del cosiddetto duello processuale. Nel confronto davanti al giudice, accusa e difesa devono essere poste in condizioni di assoluta eguaglianza: questo è chiaro e nessuno lo pone in discussione. Ma, con riferimento al processo penale, la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di ragionevolezza può ben giustificare una qualche asimmetria tra le parti, quando questa è dovuta all'esigenza di una corretta amministrazione della giustizia. Pertanto, nel processo penale, con riferimento a esempio ai rimedi, il concetto di parità tra le parti può ben trovare delle attenuazioni nel bilanciamento con altri principi pure di rango costituzionale. Del resto, la stessa sentenza n. 26 del 2007 ha ribadito che: «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà Quali sono, quindi, i principi in base ai quali la perfetta parità può essere derogata? In primo luogo, lo può essere sicuramente sull'altare del principio del *favor Nel nostro ordinamento penale vige il principio dell'*in dubio pro reo,* come abbiamo studiato tutti nei primi anni di università alla facoltà di giurisprudenza. In penale, se sussiste qualche incertezza normativa, questa deve essere sempre e comunque risolta a vantaggio dell'imputato. Nel nostro ordinamento si preferisce che magari un colpevole venga mandato assolto per quella che una volta si chiamava insufficienza di prove, piuttosto che un innocente venga condannato a una pena ingiusta. Mi sembra A questo si aggiunga che nel nostro processo penale è stato introdotto nel 2006 il concetto di ragionevole dubbio: l'imputato non può essere condannato se sussiste anche il minimo dubbio che sia colpevole. Come corollario discende un ulteriore argomento per ritenere inappellabili le sentenze di assoluzione. Infatti, come si può ritenere superato il minimo dubbio in ordine alla colpevolezza di un imputato, se un giudice, un giudice, sia esso monocratico o collegiale, magari anche adiuvato da una giuria popolare, quell'imputato in un certo grado di giudizio lo ha mandato assolto? Questo è un concetto molto chiaro negli ordinamenti di cultura anglosassone, che è stato mutuato all'interno del nostro ordinamento. Peraltro, è stato un illustrissimo giurista come il professor Tullio Padovani a suggerirlo per primo. Tale concetto è poi stato fatto proprio dalla migliore dottrina penalistica italiana. quindi, di un principio di altissima civiltà giuridica che non può essere totalmente ignorato, come invece ha fatto la pronuncia della Corte costituzionale che stiamo contestando. Ma non finisce qui. La nostra Costituzione presenta anche il principio della ragionevole durata del processo. Allora, l'inappellabilità di sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero avrebbe un effetto deflattivo, in linea con la necessità,

ha ribadito che: «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà tra accusa e difesa». Cito ora la sentenza della Corte n. 34 del 2020, che ho trovato molto opportunamente citata nel *dossier* dell'Ufficio studi. In questa sentenza la Corte, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che: «il potere di impugnazione della parte pubblica

difesa (articolo 24 della Costituzione), che ne accresce la forza di resistenza [...]». In sintesi, gli argomenti su cui si basa la sentenza n. 26 del 2007 possono essere confutati con adeguata motivazione giuridica e costituzionale e non costituiscono, quindi, un elemento ostativo all'approvazione del testo di legge oggi all'esame dell'Assemblea. Si ricorda, infine, che la sempre e pur tante volte citata sentenza della Corte n. 26 del 2007 ha bocciato la legge cosiddetta Pecorella perché non era riferita ad alcune categorie di reati, ma estesa indistintamente a tutti i processi. Proprio per superare questa censura, il testo di legge in esame prevede che l'inappellabilità riguardi non tutti i reati, ma solo quelli meno gravi, per i quali è prevista l'accettazione diretta dell'imputato. Per tutti questi motivi, argomentati motivi, argomentati e variegati, signor Presidente, la censura di illegittimità costituzionale sostenuta da alcuni partiti dell'opposizione e oggetto del presente dibattito non merita accoglimento e dovrà essere respinta.

Fondamentalmente viene posto il tema e si ritiene che l'*abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio possa portare veramente a un disfacimento del nostro panorama e del nostro ordinamento.

del tempo da dover necessariamente ridimensionarne una portata che diventa generica e quasi generalista. Il problema del reato dell'abuso d'ufficio non è dato dal fatto che è una misura considerata - come espressamente detto anche in sede di audizione da alcuni esponenti della È un reato spia per far presagire che vi sono altri reati o una modalità per cominciare a indagare al fine magari Tutti questi interventi normativi non fanno nient'altro che dimostrare che la la fattispecie prevista nel codice è un problema. Si è cercato più volte di intervenire al fine di rendere la norma più obbediente ai principi di tassatività e tipizzazione necessari nel codice penale.

Lo riconoscono anche i colleghi dell'opposizione che dicono che non ci sono tante condanne; ciò per dire che possiamo mantenere un reato perché alla fine non si è mai condannati. È questo però il problema. Se tante indagini partono e non vengono portate definitivamente alla condanna, sorge il quesito: ciò avviene perché il reato non c'è o perché esso è mal strutturato? In entrambi i casi

per esercitare qualche deviato potere. No: i reati e le fattispecie ci sono. Non per niente voi stessi dite che si può procedere eventualmente per reati anche ben più gravi, come la corruzione. Prima però di cominciare un'indagine sulla corruzione, si individuerà magari qualche elemento per non partire genericamente Quando voi scrivete della paura della firma, dite ai signori sindaci, anche ai vostri sindaci, di non aver paura perché tanto alla fine nessuno viene condannato per l'abuso d'ufficio. Dal momento però in cui si ha la notifica di un avviso di garanzia, dove si dice che si è aperto un processo, che cosa accade nei confronti di quella persona? Quella persona *in primis* è costretta a sopportare una macchina del fango terribile e inquinante nella sua vita personale, nella sua vita professionale, nella sua vita istituzionale,

la fine della sua vita politica. Vogliamo ricordare i casi di persone che sono giunte a una totale assoluzione dopo anni e nel frattempo sono state costrette a subire pesanti ripercussioni *(Applausi)* sulla propria vita politica

dell'illegittimità costituzionale, ma lasciamo che sia la Corte eventualmente a discuterne un domani. In alcuni interventi viene richiamato l'articolo 3 della Costituzione, ma non si capisce il perché:

L'altra questione che viene sollevata riguarda la possibilità per il pubblico ministero di proporre appelli nei casi di proscioglimento soltanto dei reati meno gravi. Abbiamo parlato della sentenza Pecorella e abbiamo sentito anche gli interventi dei colleghi. Non posso aggiungere molto a quello

indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale

in ordine all'esigenza di consentire a tutti i Gruppi di opposizione di avere il tempo sufficiente per poter elaborare i subemendamenti rispetto agli emendamenti presentati dal Governo sul cosiddetto premierato, che è la riforma costituzionale della nostra forma di Governo. Come è noto ai componenti della 1a Commissione, i quattro emendamenti del Governo sono arrivati sul filo di lana - diciamo così

ora noi apprendiamo che, mentre con grande fatica è stato possibile spostare il termine degli emendamenti da oggi pomeriggio alle ore domani mattina alle ore 10, su questioni non proprio banali che attengono evidentemente alla profondità del nostro ordinamento, non più tardi di un'ora fa, signor Presidente,

la norma del premierato rispetto agli emendamenti del Governo presentati ieri riguardo ai potere del *Premier* in caso di sfiducia, visto che per alcuni giuristi potrebbero essere oggetto di diverse interpretazioni. Ora, signor Presidente, noi ci troviamo nella seguente condizione: da una parte la maggioranza, come se fossimo nella carica di Balaklava, vuole portare in fondo la discussione e l'approvazione di tutti questi emendamenti, come se fossimo in una sorta di come dire palingenesi. Mille e non più mille, bisogna assolutamente fare questa riforma. Dall'altra parte, la Ministra viene a dire che gli emendamenti che ieri o, meglio, questa mattina hanno presentato potrebbero essere oggetto di ulteriore riformulazione. Noi vogliamo dire una cosa molto semplice: siccome la Costituzione non è

e venite quando finalmente avrete una proposta reale. Mi faccia dire, se lei non ha pazienza. Credo che, se ci sarà la necessità di avere tempo per valutare ulteriori eventuali emendamenti, ne prenderemo atto e daremo tutto il tempo necessario. Non mi è sembrato che ci fosse una certezza: questo volevo dire. Ad ogni dichiarazione a un giornalista, noi non possiamo stravolgere l'ordine del giorno. Se ci fossero

onorevoli colleghi, Governo, il testo che ci accingiamo a esaminare e a discutere, che poi verrà posto in votazione, ha fatto un lungo percorso ed è arrivato finalmente in Aula dopo un cammino direi molto lungo e abbastanza travagliato, non tanto nella sua vita nella Commissione dove è stato esaminato, quanto per quegli ostacoli di natura sostanziale che ha trovato sul suo percorso, quelle resistenze che sono state formulate anche a mezzo stampa, anche da parte di varie forze politiche. Da ultimo, ancor prima che prendesse le forme di un testo approvato dal Parlamento, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il testo è stato ampiamente stigmatizzato dai procuratori che hanno inaugurato i rispettivi anni giudiziari. È un provvedimento che certamente mostra una importanza e che sicuramente risponde a una richiesta che a più voci è arrivata in Parlamento, ed è arrivata a tutti i rappresentanti politici: quella, cioè, di avere una giustizia giusta. Questa è la nostra ambizione, il desiderio che cerchiamo sempre di realizzare. Una giustizia giusta vuol dire una giustizia che non ponga ostacoli all'accertamento della verità, e che soprattutto ponga al suo centro un principio di civiltà giuridica, che è poi quello al quale noi ci ispiriamo sempre, dal primo momento in cui si varcano le aule di giurisprudenza, e cioè la certezza del diritto. Il diritto deve essere certo, deve essere chiaro. La norma deve essere immediatamente percepibile e comprensibile dal cittadino comune: da quello che ha frequentato le scuole più elevate a quello che, invece, non ha potuto seguire un percorso scolastico. Entrambi, leggendo una norma di legge, devono capire qual è il comportamento vietato, qual è la condotta che si può sanzionare, qual è il divieto che il legislatore pone nel porre in essere determinate condotte. sicuramente questa certezza non riguardava l'articolo 323 del codice penale, con riferimento all'abuso d'ufficio, nella sua ultima formulazione, peraltro oggetto di ripetute modifiche da parte del legislatore. Perché erano state fatte quelle modifiche? non totale certezza del testo, per la non piena comprensione dello stesso, per la non completa attuazione di quello che è un principio che vuole che, appunto, il diritto sia certo. Ecco perché, nel tempo, esso era stato riformulato. Ma, di riformulazione in riformulazione, non si era riusciti a superare una indeterminatezza di fondo, una vaghezza nella disposizione legislativa, per la quale, sostanzialmente, ci si trovava, da operatori delle amministrazioni locali, a temere di essere accusati di abuso d'ufficio, pur nella convinzione di aver agito sempre nel giusto. di aver agito sempre nel giusto. Ovviamente, sfrondiamo il campo da quelle che sono le condotte illecite poste in essere con la consapevolezza di compiere un reato. Va da sé parliamo di quegli amministratori, tanti, numerosissimi, che invece, nel porre in essere le loro attività, si trovavano esposti a questo dubbio, a questo timore. E questo dubbio, questo timore non fugato, non affrontato correttamente, lasciato a lambire ai margini delle attività amministrative, alla fine aveva determinato la cosiddetta paralisi amministrativa, cioè il timore di firmare gli atti, di portare avanti le azioni della pubblica amministrazione, e l'inerzia, che è l'altro grande male dell'amministrazione pubblica italiana. Una pluralità di sindaci, di tutti i colori politici, sottopongono tutti lo stesso problema, rappresentano tutti lo stesso timore, dichiarano tutti di avere un'amministrazione molto spesso paralizzata dal timore di una sanzione per una condotta che può essere considerata delittuosa o ipotizzata delittuosa. Poi si fa un processo e bisogna vedere come va a finire. Ma quanti anni passano, quante risorse si impiegano e quanta è la paura. Questo, poi, ha un effetto di moltiplicazione di moltiplicazione sugli altri funzionari, sugli altri dirigenti. Basta fare caso ai dati per rendersi conto quando una norma non funziona bene. Basta guardare a quella che è la sua attuazione. Nel 2021 noi abbiamo un dato sconcertante: su 5.418 procedimenti, ben oltre il 98 per cento è andato a finire o con un'assoluzione o con un'archiviazione. Ma dietro l'assoluzione e l'archiviazione c'è ovviamente tutto un *iter* che è stato messo in atto, una fase di indagini, una fase di prima notifica, di avviso di conclusione di indagini preliminari. soprattutto, c'è un *pathos* da parte degli amministratori che non meritano, fra tutte le difficoltà nelle quali operano, di doversi confrontare con la vaghezza e l'incertezza di una norma che li espone a un pericolo,

legge in esame non è una norma bavaglio e non ha alcuna intenzione di impedire alla stampa di fare il suo dovere e rendere l'informazione ai cittadini. Anzi, direi che è una norma anti-ludibrio, anti-pubblico ludibrio.

quella pruderie - per dirla con un'espressione desueta, ma che rende secondo me assai bene il senso - di sapere determinate cose della vita privata dei soggetti coinvolti, o addirittura dei soggetti vicini ai soggetti coinvolti. Ebbene, il ministro Nordio l'ha detto chiaramente: si vuole finalmente introdurre un principio di civiltà giuridica. I soggetti terzi, che non hanno nulla a che fare con quelle indagini, con quel processo o con quell'atto, hanno diritto a non vedere violata la loro *privacy*; hanno diritto a non finire sulla carta stampata in articoli che nulla hanno a che vedere con le indagini in sé per sé, ma che coltivano quel senso un po' popolare per un'informazione che riguarda le vite private delle persone, con un certo voyerismo giudiziario che francamente non ci piace e che sicuramente non deve essere in alcun modo coltivato. Questo disegno di legge incontra certamente il favore di Italia Viva. Lo abbiamo sostenuto in Commissione e anche nei vari dibattiti pubblici. Abbiamo anche preso posizione più volte ed espresso giudizi di apprezzamento nei confronti dell'attività del ministro Nordio, perché è un provvedimento che si pone nel solco di quelle riforme che Italia Viva porta avanti e che considera necessarie per il nostro Paese. Quindi, al ministro Nordio rinnoviamo l'apprezzamento per l'attività che ha posto in essere fino adesso: certo, è un'attività che - come ho detto in premessa - ha incontrato

dalla teoria che dice che già le carriere sono separate e che sono pochissime le domande di passaggio dal ruolo inquirente a quello giudicante. Non ci interessa e non è questo il senso. Quello è un significato giuridico ancor più profondo e significa garantire il diritto del cittadino a un processo giusto, equo.

un'interpretazione autentica della legge n. 287 del 1951, quella che ha istituito in Italia le corti d'assise, e riguarda esattamente il limite di età dei giudici popolari, cioè dei componenti della giuria in corte d'assise e in corte d'assise d'appello.

del settore, ma si era creato un *vulnus* su questa normativa, perché c'era stata un'interpretazione da parte di alcuni avvocati che aveva eccepito che il superamento della soglia d'età potesse essere fatto valere anche nel corso dello svolgimento del processo. Ed era stata accolta questa eccezione, determinando la dichiarazione di nullità di alcuni processi importanti, anche delicati e particolarmente sofferti. un anno fa, durante un *question time* presentai un'interrogazione specifica al ministro Nordio sull'argomento e ho avuto il piacere di vedere

un motivo di orgoglio personale: al contrario, è motivo di grande soddisfazione perché non tutti sanno che, se questa norma non fosse stata interpretata autenticamente, anche il processo per la strage di Bologna avrebbe rischiato di essere travolto per questa eccezione e non sarebbe stato più possibile celebrarlo, perché nel frattempo erano decorsi i termini di prescrizione. *(Applausi)*. Quindi, esprimo veramente contentezza per questa norma e, in generale, con riferimento al disegno di legge

Nordio che Forza Italia considera il primo stralcio di quella grande riforma della giustizia che il nostro Paese attende e sogna da quando Forza Italia fu fondata da Silvio Berlusconi. A distanza di poco più di un anno dall'insediamento del Governo Meloni, si comincia quindi a intravedere un poderoso intervento normativo improntato ai valori del liberalismo e del garantismo giuridico. Il nostro giudizio su questo disegno di legge governativo è certamente assai positivo. Il testo che andiamo a esaminare prevede diversi interventi su vari fronti: sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado da parte del pubblico ministero, il gip collegiale, l'interrogatorio di garanzia prima delle misure di custodia cautelare in carcere e soprattutto l'abolizione dell'abuso d'ufficio e la ridefinizione del reato di traffico di influenze. L'istruttoria del disegno di legge governativo è stata particolarmente accurata sotto la guida della nostra presidente Bongiorno e ha visto la Commissione giustizia impegnata in un lungo ciclo di audizioni e poi in un serrato confronto sui diversi aspetti del provvedimento. Partiamo, Presidente dall'abolizione dell'abuso d'ufficio, che è forse il tema più caldo e che più interessa anche chi ci ascolta da casa. Come ci hanno fatto rilevare molti accademici auditi - ne abbiamo ascoltati tanti e ne cito uno fra gli altri, il professor Ambrosetti Enrico, illustre ordinario della cattedra di diritto penale dell'Università di Padova - l'attuale formulazione del reato di abuso è stata variata più volte nel corso degli anni, senza aver mai raggiunto un esito soddisfacente. Il reato di abuso è rimasto un reato a condotta evanescente, in cui il confine tra lecito e illecito è sempre stato nebuloso e generico; si è sempre prestato a interpretazioni giurisprudenziali divergenti e non uniformi, ponendosi quindi in contrasto con i principi di tassatività e legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione. A ciò si aggiunga che tale reato ha intasato gli uffici delle procure della Repubblica, impegnate in costose e inutili indagini. Qualifico inutili queste indagini perché - come ha ricordato il ministro Nordio in un'intervista del 23 giugno 2023 al «Corriere della Sera» - a fronte di migliaia di procedimenti penali aperti, solo pochissimi si sono conclusi con una condanna. Ricordava Nordio in quell'intervista che, dopo vent'anni di cambiamenti, la norma dell'abuso d'ufficio è stata un fallimento, perché su 5.000 processi sono arrivate solo nove condanne, tra l'altro tutte per reati connessi: un vero spreco di risorse. Sulla proposta di *abrogatio criminis*, l'opposizione si è divisa: Italia Viva e Azione, che pure sono forze di opposizione ma sinceramente votate alla cultura del garantismo giuridico, hanno votato a favore; mentre invece il PD e il MoVimento 5 Stelle hanno votato contro. hanno votato contro. Singolare la posizione del PD. Mentre il Gruppo parlamentare, schiacciato dalla posizione della segretaria Schlein, fa opposizione a braccetto del MoVimento 5 Stelle, i suoi amministratori locali si sono dissociati dalla posizione ufficiale del partito. Cito un intervento che ha avuto luogo in un confronto che ho avuto sulla stampa locale con l'onorevole Achille Variati, illustre esponente del PD, attuale europarlamentare, ex Sottosegretario all'interno ed ex Presidente dell'Unione delle Province italiane che, sul punto, ha affermato che era ha affermato che era e rimane assolutamente favorevole all'abrogazione di una norma scritta male, che ha generato solo problemi. Con riferimento alla posizione del Gruppo parlamentare PD, Variati ha aggiunto: «Mi dispiace molto. Credo che il PD dovrebbe imparare a parlare e ad ascoltare i suoi sindaci, che si misurano direttamente e quotidianamente con i problemi veri». Colleghi del PD, dovreste seriamente meditare su queste parole, che peraltro provengono da un vostro esponente, persona molto seria ed autorevole, perché è di tutta evidenza che la neosegretaria Elly Schlein vi sta appiattendo sulle posizioni giustizialiste e manettare del MoVimento 5 Stelle, che viceversa non perde occasione per schiaffeggiarvi su tanti temi, non ultimo il sostegno alla causa ucraina. Passiamo al tema dell'inappellabilità delle sentenze di primo grado di assoluzione da parte del pm, che è sempre stato assai caro a Forza Italia, al nostro grande presidente Silvio Berlusconi e al compianto amico e collega Nicolò Ghedini. Nel 2007 venne cancellata dalla Corte costituzionale la cosiddetta legge Pecorella, che l'aveva introdotta, e ciò è accaduto attraverso una sentenza giuridicamente lacunosa, opinabile ed intrisa di pregiudizio ideologico.

il principio viene riaffermato nel testo ora all'esame dell'Assemblea con riferimento ai reati a citazione diretta. Nel nostro processo penale vige il principio del ragionevole dubbio: l'imputato non può essere condannato, se sussiste anche il minimo dubbio che sia colpevole e come si può dunque ritenere superato il minimo dubbio in ordine alla colpevolezza di un imputato, se un giudice quell'imputato in un certo grado di giudizio lo ha mandato assolto? Questo è un concetto assai chiaro negli ordinamenti di cultura anglosassone, che è stato mutuato all'interno del nostro ordinamento, un principio di altissima civiltà giuridica che trova applicazione in questo testo di legge che oggi ci accingiamo ad approvare. Bene ha fatto quindi il ministro Nordio ad introdurlo, accogliendo tra l'altro un precedente ordine del giorno a prima firma del sottoscritto. Di grande importanza sono anche i nuovi istituti del gip collegiale e dell'interrogatorio di garanzia, prima delle misure di custodia cautelare in carcere. In questo modo si potrà significativamente rafforzare la tutela del cittadino di fronte agli abusi della carcerazione preventiva. È anche questa una riforma di straordinaria importanza. Una sottolineatura, però, ritengo di formularla al Governo: se non vogliamo veder fallire il gip collegiale, che, come ha detto tra l'altro la settimana scorsa durante il *question time* il ministro Nordio, potrà influire positivamente anche sul sovraffollamento carcerario, attenuandolo in modo significativo, si dovrà necessariamente intervenire anche con un riordino della geografia giudiziaria. Il gip collegiale non può funzionare nei piccoli tribunali, ove le incompatibilità impedirebbero la costituzione dei collegi giudicanti. Sarà inevitabile prevedere tribunali con un organico di almeno quaranta giudici, formare le sezioni gip, il tribunale della famiglia e le sezioni giudicanti specializzate previste dalla legge. Voglio sottolineare in modo particolare che nel testo di legge sono stati inseriti e approvati due nostri importanti emendamenti. Il primo riguarda l'esclusione dei brogliacci dalle informative dei aventi per oggetto intercettazioni di nominativi di soggetti terzi estranei all'inchiesta, una norma di assoluta garanzia a tutela del buon nome e dell'onorabilità dei cittadini estranei alle impugnazioni. Il secondo riguarda il divieto assoluto di intercettazioni tra avvocato e cliente. Torniamo al divieto di includere nelle informative dei pg il nome dei soggetti terzi estranei. È una norma che nei riflessi di stampa ha avuto un giudizio da parte di taluni negativo, ma che credo sia del tutto ingiustificato, in quanto in realtà tutela solo i terzi estranei, non impedisce le intercettazioni e non pregiudica i diritti di difesa, quindi siamo molto orgogliosi di aver presentato presentato quell'emendamento, che ha trovato poi il conforto e il parere favorevole del Governo. Importantissimo, a nostro giudizio, è anche il divieto assoluto di intercettazioni tra avvocato e cliente. Quest'ultimo principio pareva dovesse già essere una cosa ovvia e scontata nel nostro ordinamento, in ossequio al segreto professionale, ed invece è ancora violato con sorprendente disinvoltura. La cronaca quotidiana, peraltro, ci ricorda quanto questo nostro emendamento fosse assolutamente provvidenziale e necessario di fronte ad evidenti abusi delle procure. Pochi giorni fa credo che tutti ci siamo sdegnati quando abbiamo visto che sono state divulgate le intercettazioni registrate tra il legale della Pifferi (quella sventurata madre omicida) e le psicologhe del carcere di Milano ove la Pifferi è reclusa,

Mi viene in mente un'altra vicenda di cui si è occupata la stampa, quella dell'avvocato Francesco Perli, noto amministrativista che assisteva l'Ilva davanti al Consiglio di Stato di cui la stampa in passato ha parlato a lungo. Il legale è stato intercettato per mesi mentre discuteva la linea difensiva con i propri assistiti, addirittura mentre si svolgeva l'incidente probatorio, e le intercettazioni sono state usate nel processo come prova a suo carico. C'è quindi davvero bisogno di vietare definitivamente questi clamorosi abusi. Il segreto professionale dell'avvocato ha rango primario e non può essere violato in modo così palese, addirittura per condizionare i processi in corso. Ora, con l'approvazione del nostro emendamento, finalmente la questione sarà chiarita una volta per tutte. Tuttavia, signor vice ministro Sisto, al testo mancano due aspetti sui quali conto di tornare: la previsione di un illecito disciplinare specifico a carico del magistrato che viola il divieto e un elenco di udienze di cui sono titolari gli avvocati, che mai e poi mai possono essere oggetto di intercettazione, quali che siano i motivi. In conclusione del mio intervento, desidero rimarcare un aspetto molto positivo, politico e metodologico, del ministro Nordio. In genere si accusa il Governo (non solo quello presieduto da Giorgia Meloni, ma in generale i Governi che si sono succeduti negli anni) di schiacciare Camera e Senato e di trattarli come meri passacarte, chiamati solo a ratificare i decreti-legge.

(lo sottolineo con grande piacere): ne fanno prova gli importanti emendamenti citati e accolti all'interno del presente disegno di legge, nel quale sono anche stati accolti emendamenti dell'opposizione (penso a quello molto importante che elimina, per gli avvocati di fiducia, l'obbligo di ottenere un nuovo mandato dal cliente per l'impugnazione; è un fatto molto tecnico che riguarda la categoria degli avvocati, ma che è stato molto apprezzato). Mi sembra che il tempo stia per scadere: in conclusione, vorrei ringraziare la presidente Bongiorno per l'eccellente lavoro che è stato svolto in Commissione, gli uffici e l'ufficio studi. particolare al qui presente vice ministro Sisto - che questa è solo la prima delle battaglie sulla giustizia; so che con lui sfondo una porta aperta, ma il tema della separazione delle carriere dei giudici è pregnante e qualificante, soprattutto per il nostro partito. Pertanto, pur comprendendo che non può andare di pari passo con la riforma del premierato,

Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, oggi discutiamo della riforma della giustizia, fortemente voluta e rivendicata dal Governo Meloni. riforma dimostra esattamente come questo Governo ignori totalmente quello che chiedono le persone e si muova solo in un'unica direzione: quella di difendere gli interessi corporativi dei soliti noti, cioè potenti e colletti bianchi.

esattamente il contrario di quello che prevede la riforma Nordio, che va inserita in un contesto che, con provvedimenti disseminati un po' qui e un po' là, restituisce un quadro d'insieme davvero preoccupante, per cui la giustizia italiana diventa drammaticamente lenta, incerta e ingiusta. I cittadini chiedono una giustizia veloce e per suo tramite, signora Presidente, vorrei che il Governo spiegasse ai cittadini italiani come velocizzerebbe un procedimento, per esempio, far passare la decisione sulla custodia cautelare da un solo magistrato in capo a tre magistrati. In pratica, quello che faceva prima un solo magistrato, oggi lo devono fare in tre. A occhio e croce il tempo si triplica per ogni decisione e non credo che serva un disegnino esplicativo per comprenderlo, a meno che il ministro Nordio non intenda e non preveda che i cinque giorni di preavviso da dare all'indagato prima dell'applicazione della misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione non assolvano allo scopo di accelerare i processi. processi. Effettivamente infatti dare all'indagato la possibilità di inquinare le prove o di rendersi irreperibile indubbiamente velocizzerebbe i tempi della giustizia, perché non ci sarebbe nessun processo da celebrare. Se poi registriamo che, da quando questo Governo è in carica, non è stato destinato un solo euro all'incremento del personale, unica e vera risposta all'ingolfamento delle procure, mi sembra evidente che questo Governo non abbia nessun interesse a velocizzare proprio un bel niente. E mi fa sorridere vedere il ministro Nordio compiacersi per le 4.000 unità di personale incrementate o per l'approssimarsi dei tre concorsi per circa 1.300 magistrati ordinari. Vorrei ricordare al Ministro, sempre per suo tramite, Presidente, che il suo è solo un maldestro tentativo di intestarsi il risultato del piano di assunzioni di ben 15.000 unità, varato a partire dal 2018 dal Governo Conte I. *(Applausi)*. Questa è l'unica vera riforma per una giustizia veloce, come chiesto dai cittadini. Passiamo al secondo punto. I cittadini chiedono una giustizia certa. Anche qui, Presidente, sempre per suo tramite, vorrei che il Governo illustrasse ai cittadini e a noi in questo Senato come si risponda in questo modo all'esigenza di una giustizia che punisca con certezza chi compie un reato come violenza, ricettazione o truffa. truffa. In questa riforma si prevede infatti che venga impedito ai pubblici ministeri di ricorrere in appello in caso di assoluzione in primo grado. Vorrei solamente ricordarvi che la giustizia italiana prevede tre gradi di giudizio; quindi di interrompere un procedimento dopo il primo grado, replicando l'impianto della legge Pecorella, che, come ricordato, è stata dichiarata incostituzionale, altera gravemente le condizioni di parità tra imputato e pubblico ministero. Se a questo aggiungiamo il ritorno della prescrizione, il cerchio si chiude. L'imputato più facoltoso potrà permettersi infatti stuoli di avvocati bravissimi a trovare ogni minimo cavillo per dilatare i tempi e far sì che la giustizia non faccia il proprio corso. Il risultato evidente, perseguito da questo Governo, è la certezza, sì, però dell'impunità. Il ministro Nordio si guarda naturalmente bene dal confronto con i Governi Conte: non sia mai che i cittadini si accorgano della differenza tra chi si è adoperato per una giustizia equa e chi riesuma i baluardi della giustizia classista, tanto cara alla maggioranza che si nasconde dietro il garantismo mentre mira a garantire l'impunità dei reati tra i più odiosi e i più dannosi per la collettività. Veniamo così al terzo punto. Sì, i cittadini chiedono una giustizia giusta e, sempre per suo tramite, Presidente, vorrei chiedere al Governo come cancellare l'abuso d'ufficio e limitare il reato di traffico di influenze illecite garantirebbe i cittadini da condotte fortemente lesive della legalità e del bene collettivo. Voglio fare qualche esempio. L'abuso d'ufficio è la porta da cui s'infiltrano malaffare e mafie per influenzare la pubblica amministrazione. Si pensi al sacco di Palermo e ai permessi di costruzione rilasciati nottetempo per zone non edificabili o soggette a vincoli. Senza arrivare alle mafie, si pensi agli abusi nella sanità, con i medici pubblici che dirottano i pazienti verso strutture private; si pensi ai concorsi truccati a favore di candidati raccomandati, com'è successo recentemente proprio nel concorso in magistratura. Durante la prova - rinfresco un po' la memoria a chi forse non si è accorto di quello che è successo - un candidato ha tentato di rendere riconoscibile, con segni di identificazione, il proprio tema, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo sul proprio scritto. Per errore, il messaggio è stato inviato a un altro commissario.

Come si pensa di proteggere la cosa pubblica indebolendo e cancellando, uno ad uno, i presidi di legalità che avevamo posto a difesa dei cittadini nel Governo Conte I con la cosiddetta spazzacorrotti? Colpendo gli strumenti più efficaci che hanno i magistrati, come le intercettazioni? Tra l'altro, il ministro Nordio è davvero sfortunato, perché non fa in tempo ad attaccare questo presidio di intercettazioni al servizio della magistratura, che viene arrestato Matteo Messina Denaro e il procuratore De Lucia sottolinea senza alcun indugio che senza le intercettazioni questo risultato non si sarebbe mai potuto raggiungere. *(Applausi)*. In definitiva, questa riforma va esattamente dalla parte opposta di quello che chiedono i cittadini: al posto di una giustizia veloce, certa e giusta, rifilerete agli italiani tempi dilatati, certezza dell'impunità e una giustizia classista; una giustizia dai guanti di velluto con corrotti, corruttori e colletti bianchi, che lascerà sempre più soli e indifesi i cittadini alla mercé del potente di turno.

sulla norma principe, quella che andrà ad abrogare l'abuso d'ufficio, ma vorrei fare una considerazione sull'intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, che oggi non è soltanto obsoleto, ma è divenuto anche un campo di manovra politico per un'area di pensiero che ha provocato un unico certo effetto, e lo hanno ricordato alcuni dei colleghi prima di me: la diminuzione dell'efficacia dell'azione amministrativa proprio tra i funzionari più ligi al dovere, che evidentemente di patire conseguenze dovute a norme che si prestano a una diversificata e molto discrezionale applicazione.

È assurto addirittura, da parte di una certa area dottrinaria e giudiziaria, alla qualificazione di reato spia, secondo modelli che definisco esplorativi o predittivi tipici di sistemi inquisitori sovietico-cubani, per non parlare del traffico di influenze illecite. Chi si contrappone oggi a questa riforma ha abusato del concetto di reato spia, che per lo più è affine alla materia dell'antimafia, che lo considera nella disciplina amministrativa dell'informazione antimafia interdittiva una condotta che riflette in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale e intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso.

L'accusa infamante appare dunque un ultimo appiglio degli irriducibili, i quali probabilmente rappresentano a loro volta il timore di coloro che temono una perdita nella loro personale non eccelsa azione investigativa o giudiziaria o l'ulteriore paura di dover iniziare a confrontarsi con l'esigenza di più puntuali elementi indiziari e di prova rispetto a ciò che hanno solo astrattamente teorizzato attraverso l'abuso d'ufficio, fino ad oggi. Una certa area politica, colta da ciclico tripudio di fanatismo politico-giudiziario contro ogni figura di amministratore pubblico, ha accolto questa istanza e ha inteso farne a più riprese la bandiera del proprio sadismo giudiziale. La verità è che, in ragione di una guerra santa ai colletti bianchi, molti ambiti della nostra azione preventiva contro la vera criminalità, quella scomoda, quella di strada, sono passati nelle mani di coraggiosi magistrati ai quali è stata fino ad oggi preclusa dalle correnti della magistratura, guarda caso, una dignitosa e meritata carriera. Gli altri invece hanno alimentato alcune maxi-inchieste, con con quella che potrebbe essere definita una surrettizia applicazione dei criteri prioritari nella trattazione degli affari penali, preferendo fare indagini sui colletti bianchi, tralasciando tutta una serie di fattacci che magari non fanno *curriculum* giornalistico trascurando quindi di perseguire i reati che colpiscono invece la gente comune. Di certo e nella quasi totalità dei casi il colletto bianco è un soggetto ideologicamente comodo da colpire: non sbarca a Pozzallo o a Lampedusa, non spara, non non minaccia e non fa parte di gruppi armati organizzati; in qualche caso, forse alimenta sistemi criminali (certo, a volte), ma si tratta di una caccia alle streghe pulita, che ha il vantaggio, attraverso la rilevante ricaduta mediatica del fatto, di costringere il soggetto, anche a causa della troppo frequente diffusione dei contenuti di conversazioni intercettate, all'abbandono in perpetuo per ragioni di opportunità, quando non per obbligo di legge, di posti di rilievo politico-amministrativo, di cui guarda caso poi possono beneficiare altri, con evidenti effetti nella competizione politica. Non abbiamo infatti mai assistito a manifestazioni di solidarietà verso imputati assolti dopo anni di gogna mediatica; abbiamo assistito invece all'indignazione di alcuni magistrati, anche del CSM, per le riprese video effettuate in luogo pubblico a una loro collega che manifestava contro le politiche migratorie del Governo e di Matteo Salvini.

sapiente costruzione mediatica, che ha avuto l'effetto di infangare l'immagine del Paese a livello internazionale. Il disegno di legge Nordio agisce rispetto alla necessità di disinnescare alcune fra le più frequenti conseguenze dell'azione processuale penale dettata dalla virulenza della capacità intrusiva e distorta dell'uso del mezzo informativo, che può costituire una delle fonti più appetibili di *scoop* mediatico, utile a ragguagliare il lettore o lo spettatore su vicissitudini che non erroneamente sono state definite un'anticipazione della pena sotto forma di gogna mediatica. L'informazione in stampa, non per sua colpa, è ormai divenuta un elemento altamente delegittimante delle istituzioni, sul quale poggia e si alimenta una consistente porzione del comune sentire della società contemporanea. Ciò accade ancor di più quando l'origine di queste informazioni siano i contenuti sempre più invasivi delle attività di ascolto investigativo, attraverso strumenti di captazione o intrusivi. Non possiamo che concludere esprimendo la nostra posizione a favore delle modifiche codicistiche contenute in questo testo, che prende non a caso il nome del ministro Nordio, appunto al Ministro - stimoli una lotta più incisiva alle vere aggressioni al nostro sistema amministrativo, dismettendo atteggiamenti prevenuti verso coloro che hanno scelto di servire le istituzioni pubbliche e lo fanno con dignità,

molto modesto rispetto alle ambizioni sbandierate e denunciate. È molto modesto perché è un provvedimento che incide poco o forse nulla sul piano dell'efficienza, della velocizzazione dei processi e del miglioramento del nostro sistema e del nostro apparato.

giustizia, e lo fa anche con tante contraddizioni, tra i principi che vengono sbandierati e si intendono tutelare e quello che concretamente

Il caposaldo attorno al quale sono state costruite l'immagine e la comunicazione mediatica di questo provvedimento è il tema dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, che noi abbiamo ritenuto e riteniamo un grave errore. Non solo noi, per la verità, perché, se qualcuno avesse voglia di leggere o ascoltare le audizioni che abbiamo fatto, nel corso della lunga istruttoria che ha preceduto l'arrivo in Aula di questo provvedimento,

l'abuso d'ufficio, com'è stato detto e ricordato da quasi tutti gli auditi, è una norma di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, senza la quale si rischiano grandi buchi di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione. Questa norma non si rivolge solo ai sindaci, ma colpisce gli colpisce gli abusi di potere di tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione, tant'è vero che le statistiche dicono che per cento delle sentenze definitive di condanna per abuso d'ufficio non riguardano i sindaci, ma altri esponenti della pubblica amministrazione, in particolare

dipendenti o consulenti esterni di aziende pubbliche o di enti territoriali, direttori di carcere, presidi, professori, ricercatori universitari, medici, direttori di strutture sanitarie o altri esercenti professioni sanitarie, esponenti delle forze dell'ordine o giudici. La norma si applica, cioè, a tutti gli esponenti della pubblica amministrazione e non solo ai sindaci. Dopodiché, siccome utilizzate come pretesto sempre quello dei sindaci, voglio essere abbastanza chiaro su questo. Conosciamo bene i problemi dei sindaci, perché coi nostri sindaci ci parliamo e condividiamo le preoccupazioni che hanno sempre espresso in merito al rischio di essere indagati per reati che poi si scopre essere non sussistenti o infondati. Conosciamo bene queste preoccupazioni e le condividiamo, perché sappiamo bene che l'amministratore pubblico è soggetto al controllo della pubblica opinione e la reputazione per un amministratore pubblico è il bene più prezioso. I sindaci sono quindi effettivamente soggetti deboli da questo punto di vista, perché nel momento in cui vengono sottoposti a un'inchiesta,

che non si possono affrontare con una scelta draconiana, come l'abrogazione *tout court* di una norma che si applica a tutta la pubblica amministrazione e rischia di aprire buchi normativi di tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione che non sono minimamente coperti da altre norme.

Non possiamo solo affidarci alle richieste, pur legittime, di un sindaco, senza porci il problema dell'impatto che hanno le nostre scelte su materie così delicate come il codice penale. Questo è il punto, perché se l'impatto di quelle scelte,

da qui, ricordando che, proprio per andare incontro alle esigenze che hanno formulato molti amministratori locali, tra cui tanti del Partito Democratico, noi già nel 2020 eravamo intervenuti per l'ennesima volta - è vero, perché purtroppo sull'abuso d'ufficio si è intervenuti tante volte in questi anni, non dobbiamo nascondercelo - con una riformulazione dell'abuso d'ufficio, che, a detta di molti osservatori, ne aveva risolto il principale problema, cioè aveva tolto il controllo di legalità sull'abuso della pubblica amministrazione, quando quel presunto abuso coinvolgeva il potere discrezionale, cioè a dirsi il potere politico della pubblica amministrazione. Siccome l'accusa e il problema che erano stati sollevati stavano nel fatto che, attraverso il reato di abuso d'ufficio, si rischiava di attribuire alla magistratura il controllo politico sulle scelte della pubblica amministrazione, siamo intervenuti e abbiamo tolto quella parte: oggi parte: oggi il reato di abuso d'ufficio si applica solamente quando le norme che si assumono violate da un esponente della pubblica amministrazione sono a carattere vincolato, cioè che non danno alcuna discrezionalità e alcuna scelta di natura politica al pubblico amministratore. Abbiamo quindi ridotto il perimetro della norma e questo ha prodotto degli effetti. Infatti, anche qui, cari colleghi, non è possibile continuare a sentir dire che la norma dell'abuso d'ufficio produce una serie di guasti che non si è mai riusciti a sanare, perché, da quando abbiamo cambiato nel 2020 quella norma, il numero di indagini e poi di archiviazioni e di condanne si è sensibilmente abbassato, il che significa che il tentativo che è stato fatto di circoscrivere l'applicabilità e la portata di quella norma ha funzionato. Quel tentativo ha funzionato e quindi oggi l'idea di intervenire nuovamente con questa scelta così estrema di abrogare il reato di abuso d'ufficio senza neanche neanche fare una verifica e chiedersi se la modifica del 2020 abbia avuto un impatto sull'ordinamento è un modo di legiferare che riteniamo profondamente sbagliato. quando si fanno le riforme, prima di fare cambiamenti ulteriori, si verifica se quelle precedenti hanno funzionato, quand'anche siano state fatte da un'altra maggioranza politica, altrimenti

che sono tante le archiviazioni e le assoluzioni rispetto alle indagini aperte in tema di abuso d'ufficio. È vero: sono tante le archiviazioni, per cui più dell'85 per cento dei procedimenti viene archiviato.

nella giustizia, continuerà a denunciare, quando si sentirà abusato dal potere della pubblica amministrazione. Continuerà a farlo e continueranno ad aprirsi indagini che, nella stragrande maggioranza dei casi (come capita adesso), verranno archiviate, perché il filtro della magistratura funziona. Le indagini vengono archiviate, quando non sono fondate le denunce. Ma cosa succederà, quando arriveranno queste denunce e non ci sarà più l'abuso d'ufficio? Secondo voi, cosa farà un magistrato al quale viene sottoposta una denuncia perché un pubblico amministratore o qualche altro esponente della pubblica amministrazione hanno dato un permesso che non doveva essere dato o non hanno concesso una licenza che doveva essere data? Archivierà oppure proverà a indagare e a verificare se per caso dietro non ci sia qualcosa di più di un abuso d'ufficio e quindi iscriverà

ma lo dicono fior di avvocati insospettabili di avere simpatie per la sinistra o di essere giustizialisti, visto che l'accusa che ci fate sempre è di difendere l'abuso ufficio perché siamo giustizialisti. L'avvocato Franco Coppi dice che abrogare l'abuso d'ufficio è una boiata e una stupidaggine, perché a quel punto i magistrati indagheranno per reati più gravi.

stato un *boomerang* per gli amministratori. Non sarà la soluzione ai loro problemi, ma un *boomerang*, quindi è un grave errore anche da questo punto di vista. Dicevo che è una norma di chiusura dei reati contro la pubblica amministrazione. Qualcuno ha detto che si tratta di

Ma il punto non è questo. Forse non avete capito cosa significa reato spia. Il punto è - come ci ha detto il procuratore nazionale antimafia Melillo, che noi stimiamo - che quei reati di abuso d'ufficio

venir meno la possibilità di partire da lì, si rischia - questo dicono i magistrati che stanno sul campo contro la criminalità organizzata - di impedire di scoprire anche malaffari molto più grandi che ci stanno dietro.

quanto ciò sia ridicolo, utilizzo le parole di un altro grande giurista, che è un campione del garantismo, uno dei degli esponenti principali del filone garantista che è tanto presente nel nostro Paese. Mi riferisco al professor Tullio Padovani, Tullio Padovani, accademico dei Lincei e giurista stimatissimo soprattutto dagli ultragarantisti. Ebbene, il professor Padovani afferma che l'abolizione dell'abuso d'ufficio è una scelta assurda, improponibile si verrà a creare un buco nel quale si insinua un potere sottratto a ogni controllo di legalità. In sostanza, In sostanza, il pubblico ufficiale rimarrà titolare esclusivo di una potestà di cui non deve rendere conto a nessuno. Saremmo in uno Stato premoderno,

Voi state mettendo in discussione lo Stato di diritto, perché è proprio della separazione dei poteri consentire il controllo sull'esercizio della pubblica amministrazione da parte dei giudici e dei magistrati. Voi state facendo l'esatto contrario. Siamo noi che stiamo difendendo i principi liberali dello Stato di diritto. È l'esatto contrario di quello che continuate a dire e ve lo dicono anche giuristi liberali e garantisti come Tullio Padovani. Cito anche un altro avvocato non sospetto di simpatie con il centrosinistra, perché anzi è stato un noto esponente del centrodestra, l'avvocato Gaetano Pecorella, il quale, intervistato sul tema dell'abuso ufficio, ha detto: «tra i processi per abuso d'ufficio andrebbero consentiti quelli relativi ai conflitti di interesse: qui il reato è meno vago, rimanda a circostanze ben determinate. Sarebbe meglio non dare l'impressione di voler sdoganare qualsiasi condotta ora che c'è da gestire il PNRR. Scrivere le leggi è cosa troppo seria perché la si possa lasciare al legislatore, dicono. Senza arrivare a tanto, meglio evitare svarioni». Voi non vi limitate ad abrogare la parte della norma sull'abuso d'ufficio che interessa ai sindaci, ma eliminate anche la parte successiva, quella che impone al pubblico funzionario che ha un conflitto di interessi nel provvedimento che deve prendere di astenersi, perché altrimenti commette un reato. Togliete perfino questo che non c'entra nulla con le motivazioni che continuate ad addurre sui sindaci: anche questo è conflitto di interessi. Perfino l'avvocato Gaetano Pecorella vi dice che è una stupidaggine colossale togliere perfino questo livello di presidio di legalità su una materia così importante e delicata e anche su una parte della norma che voi volete togliere.

imporrebbe il conflitto di interessi. È stato eccepito che in realtà tale Convenzione suggerisce, non impone, agli Stati di prevedere il conflitto d'interessi. Voi, però, sapete che c'è una direttiva in corso di approvazione

una norma che punisce l'abuso d'ufficio. Se questa norma entrerà in vigore, la nostra normativa nazionale con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio entrerà in diretto contrasto con la normativa europea. Quindi, sarete costretti a tornare sui vostri passi. C'è però qualcuno che sostiene - e io penso che abbia ragione, la cosa non è mai stata indagata a fondo - che comunque con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio noi siamo già in contrasto con la normativa europea, quantomeno sotto il profilo del fatto che viene eliminato anche il peculato per distrazione internazionale, che invece è obbligatorio secondo le convenzioni internazionali. E questo ci pone in diretto contrasto con le convenzioni europee, per cui siamo anche in contrasto e in violazione con le normative europee.

poco tassativa, molto generica e su questo possiamo essere abbastanza d'accordo. Tuttavia, se si interviene su un reato così delicato, bisogna farlo bene. Il bene. Il reato di traffico di influenze è stato introdotto nel nostro ordinamento per combattere la corruzione, cioè il reato che colpisce i cosiddetti faccendieri, i mediatori tra il privato e il pubblico ufficiale, che molto spesso sono alla base degli episodi di corruzione. Colpendo i mediatori, si anticipa la lotta alla corruzione, perché si colpisce il soggetto che porta il privato a diretto contatto col pubblico ufficiale per il patto corruttivo. quando si tocca questa fattispecie si deve stare molto attenti, perché è molto importante per anticipare la lotta alla corruzione. Voi lo avete fatto in modo abbastanza limitato, ma con alcuni gravi errori. Il primo degli errori è il fatto che avete tolto dalla fattispecie del traffico di influenze la possibilità che il mediatore venga ricompensato con utilità di qualunque genere. Avete previsto solo l'utilità economica, disallineando così la fattispecie di traffico influenze dalla fattispecie di corruzione, in cui invece qualunque utilità è oggetto del patto corruttivo. Questo è quindi un disallineamento. Soprattutto, però, avete tolto dalla fattispecie la possibilità che il mediatore, il faccendiere, quello che si fa dare soldi per andare a parlare col pubblico ufficiale,

se io privato cittadino do 15.000 euro a un faccendiere che si propone di andare a parlare con il suo amico, direttore tecnico di un Comune, affinché questo mi rilasci un permesso di costruire in una zona sismica, dove io non avrei alcun potere di costruire, ora né il faccendiere né il tecnico, che rilasciasse il permesso abusivo illegittimo, sarebbero più puniti.

Questo è l'esito delle vostre scelte in tale campo. Non mi pare francamente che si vada nella direzione dell'interesse e della tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione e della corruzione.

sotto il profilo dell'impatto che avranno sul nostro ordinamento giuridico. Sono però anch'essi molto criticabili; non così critici, ma molto criticabili. Avete previsto che le misure cautelari, in particolare la misura della custodia cautelare possa essere emessa soltanto da un collegio.

Quindi, in linea di principio, va tutto bene. C'è però un piccolo particolare che vi hanno detto tutti e che anche voi sapete benissimo; il fatto cioè che non ci sono i giudici

l'interrogatorio di garanzia va sempre bene e noi da questo punto di vista non abbiamo nulla da dire. Diciamo però che anche questa è una norma che avrà una portata pratica risibile. in conclusione, il divieto di appello delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri per alcune categorie di reati. noi in linea di principio non siamo ostili a una previsione che riduca l'appellabilità anche da parte dei pubblici ministeri. Sappiamo

che prevedeva esattamente una limitazione dell'impugnazione da parte dei pubblici ministeri, ma parallelamente una rivisitazione delle impugnazioni di tutte le parti. Ci avete risposto di no

Ho sentito prima il collega Zanettin sostenere che questo è uno dei motivi che hanno suggerito tale scelta. Ma noi sappiamo benissimo che le impugnazioni da parte dei pubblici ministeri sono nell'ordine di pochi punti percentuali sul totale delle impugnazioni. Quindi,

riteniamo che il provvedimento in discussione sia per molti aspetti sbagliato e pericoloso e non produrrà alcun risultato utile sulla durata, sull'efficienza, sulla qualità dei processi in Italia. Quindi, noi voteremo convintamente contro

Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, mi permetta di intervenire su alcuni punti che hanno stretta afferenza con ciò che oggi trattiamo. Il caso di Ilaria Salis sta dimostrando quanto sia importante la diplomazia e l'azione degli Stati nella trattazione di tematiche afferenti alla giustizia. Da padre, capisco lo struggimento del signor Salis, ma da uomo delle istituzioni - come tutti noi in quest'Aula dovremmo essere - non posso che sostenere, al di là delle bandiere di partito, il Governo italiano e la sua azione diplomatica, che sarà ferma e decisa nel rispetto dei diritti fondamentali, sia chiaro, Presidente - proprio perché parliamo di giustizia, non può entrare a gamba tesa sulle decisioni della magistratura di un'altra Nazione europea. il ministro Nordio, profondo conoscitore del diritto e dei meccanismi giudiziari, essendo stato magistrato, che sta seguendo il caso con il ministro Tajani, così come sta seguendo il tema della misura cautelare e della difesa della dignità della persona. Dignità della persona e misure cautelari sono argomenti che entrano direttamente in questa riforma e fa specie che spesso coloro, che dai banchi dell'opposizione strepitano e si lasciano andare a critiche demagogiche, siano gli stessi che hanno governato l'Italia e la giustizia esprimendo propri Ministri per dieci anni. *(Applausi)*. Fa specie proprio perché sulla tutela degli italiani all'estero questo Governo, in un anno e quasi un mese, ha ottenuto risultati molto importanti: la scarcerazione di Patrick Zaki e la liberazione di Alessia Piperno sono risultati ottenuti grazie a un'azione diplomatica sottotraccia. L'auspicio - penso condiviso da tutta l'Assemblea - è di far lavorare la nostra diplomazia per consentire le migliori garanzie processuali e di custodia cautelare possibili Ilaria Salis, così come per ogni altro detenuto italiano in un'altra Nazione, e sono purtroppo centinaia. Un altro nome che deve risuonare in quest'Aula è quello di Beniamino Zuncheddu, il simbolo vivente dei tragici errori della giustizia *(Applausi)*, in grado di condizionare per oltre trent'anni la vita di un uomo. Questo deve portarci a riflettere seriamente sulla giustizia, sulla responsabilità dei magistrati, sugli errori giudiziari, sulla carcerazione e sulla situazione degli istituti di pena. Il numero dei suicidi allarma il Governo, che ha ereditato una situazione di sovraffollamento e di profondi *deficit* nell'edilizia penitenziaria. Il sovraffollamento, tra le varie cause, dipende anche dal numero di carceri disponibili, che devono essere aumentate. Sempre sul sovraffollamento incide la carcerazione preventiva che per molti imputati, poi assolti, si è rivelata ingiustificata, con un danno enorme. La nostra riforma, devolvendo a tre giudici e previo interrogatorio per l'applicazione della custodia cautelare, ridurrà questo fenomeno che confligge con la presunzione di innocenza dettata dalla Costituzione e dall'Unione europea. temi nodali, signor Presidente. L'inefficienza della macchina giudiziaria, unita a ciò che ho elencato, è uno degli ostacoli principali allo sviluppo della Nazione. Sin dal suo insediamento, dunque, il Governo ha messo a terra una serie di interventi in materia di giustizia. Tra i più significativi in termini politici si annovera, ad esempio, l'immediato intervento per salvare l'istituto dell'ergastolo ostativo, per renderlo conforme alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e dalla CEDU; tentativo peraltro fallito dalle precedenti variopinte maggioranze, che avevano partorito una norma che avrebbe completamente svuotato il senso dello strumento. Oggi ci apprestiamo ad approvare un altro tassello della riforma annunciata, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio; le modifiche al cosiddetto traffico di influenze illecite, che viene ridimensionato; la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni non penalmente rilevanti e la previsione di limiti alla possibilità per il pubblico ministero di ricorrere in appello. Il disegno esalta la volontà politica del Governo di procedere sulla strada delle riforme, in particolare di quella della giustizia, anche tramite l'assunzione di nuovi magistrati, con i bandi di nuovi concorsi e da subito 250 posti. Ma andiamo all'abuso d'ufficio. È un dato di fatto, colleghi, che la genericità dell'attuale formulazione dell'articolo 323 del codice penale ne ha determinato un'applicazione inefficace. Parlano i dati, e la matematica non è un'opinione. Oltre l'85 per cento dei procedimenti penali aperti per abuso d'ufficio è stato archiviato. Solo nel 2021, su 5.418 procedimenti ben 4.613 sono stati archiviati su richiesta del pubblico ministero, all'esito delle indagini preliminari. Il reato di abuso d'ufficio non è servito per debellare comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione; ma è stato usato, al contrario, per condizionarne l'azione. L'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale è stata quindi una scelta drastica,

Chiedetelo ai consiglieri comunali, agli assessori e ai sindaci che cosa vuol dire essere raggiunto da un avviso di garanzia e doversi dimettere per resistere alla gogna mediatica, per poi negli anni essere assolto. Nel frattempo una vita, una carriera politica e il voto di tanti cittadini vengono massacrati dai giornalisti e spesso anche da un'opposizione di parte. *(Applausi)*. La nuova previsione legislativa intende proseguire sulle linee tracciate dalla giurisprudenza, intervenuta per superare l'indeterminatezza della disposizione e tipizzare così la fattispecie di reato. Peraltro, è previsto anche l'aumento delle pene. Oggi reputazione e dignità, per quanto garantite dal principio costituzionale della presunzione di innocenza, difficilmente riescono a essere riacquistate dopo campagne giornalistiche denigratorie.

di altri reati, in quanto proprio la Costituzione, con la previsione del principio di legalità *ex* articolo 25, insegna che un reato o esiste o non esiste.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 Oggi a maggior ragione, in quest'epoca di sfide, con i progetti legati al PNRR, non possiamo permetterci blocchi che penalizzino la realizzazione delle opere pubbliche. Per quanto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 La pubblicazione di un'intercettazione potrà avvenire soltanto dopo che il giudice ne ha fatto menzione tra le motivazioni di un provvedimento, o perché così è emerso in sede di dibattimento. In più, si tutelano la posizione e l'anonimato di terzi soggetti, diversi dalle parti e quindi non partecipi della vicenda penale. Troppo spesso, Presidente, la gente viene tirata dentro per i capelli in situazioni processuali, senza avere alcun collegamento con i reati contestati nessuna scusa da parte di nessuno. Mi pare che sia una norma di civiltà minima, nonché ulteriore garanzia che rafforza la concreta applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza. Signor chiaro che le intercettazioni sono e rimangono uno strumento indispensabile per le indagini sui reati gravi; ma se ne è fatto un uso eccessivo, sproporzionato nel numero e dai costi elevatissimi; a volte, sono sfuggite al controllo. L'interrogatorio preventivo, poi, nel disegno di legge prevede di poter procedere all'adozione della custodia cautelare in carcere, previo esperimento dell'interrogatorio, secondo le modalità previste dal codice stesso, fatte salve eventuali circostanze gravi o la flagranza di reati: quindi, secondo il principio di contraddittorio tra le parti. Peraltro, anche il termine di cinque giorni rientra nella migliore esplicazione del diritto alla difesa e non implica, in alcuna maniera, che possa mai favorirsi l'indagato a discapito delle esigenze di giustizia, poiché, ad esempio, il termine viene meno in caso di pericolo di fuga. Con la riforma dell'articolo 593 del codice penale è previsto poi il divieto per il pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento in primo grado per reati meno gravi, per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. nelle ipotesi di reati meno gravi, chi verrà prosciolto in primo grado non correrà più il rischio di vedersi condannato in secondo grado, in quanto il pubblico ministero non potrà proporre l'appello. Il fatto, poi, che tale divieto sia comunque limitato esclude che possano assumersi i profili di incostituzionalità, come è accaduto con la cosiddetta legge Pecorella. come già dichiarato, il provvedimento in esame è solo un primo passo verso una riforma integrale della giustizia, volta a migliorare il funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono coinvolte. Stiamo lavorando per un sistema più garantista. Le riforme in materia di giustizia le facciamo perché necessarie, perché le avevamo promesse in campagna elettorale e perché gli italiani le vogliono fortemente, e non per resistere a presunti attacchi della magistratura. *(Applausi)*.

i roboanti annunci della campagna elettorale di un anno e mezzo fa e le continue polemiche degli esponenti dei partiti di maggioranza facevano pensare che in quest'Aula sarebbe arrivata una riforma strutturale della giustizia e non una riforma gridata. legge oggi in discussione, invece, è un provvedimento parziale, un piccolo tassello di un mosaico che conferma quanto già abbiamo denunciato in più occasioni: assenza di visione rispetto ai principali problemi dell'amministrazione della giustizia, primo fra tutti l'assenza di risorse di personale, e una volontà chiara, precisa, di smantellare pezzi importanti dell'ordinamento giudiziario, mettendo a rischio il lavoro degli organi inquirenti. Signor Presidente, vi è grande preoccupazione per i provvedimenti che questa maggioranza intende portare avanti. Questo disegno di legge in poche pagine rischia di smantellare alcuni capisaldi della lotta alla corruzione - l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze poi nuove norme sulle intercettazioni, di cui non si comprende la logica e che rischiano di andare in conflitto con il principio di trasparenza degli atti e con il diritto all'informazione. Ancora, in questo disegno di legge si introduce la riduzione della possibilità di fare appello per il pubblico ministero e si modifica la composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere: una norma che sembra ispirata da semplice populismo, vista l'assenza di risorse e di personale, che rendono impossibile allargare la composizione dei collegi giudicanti, ma che rischia, allo stesso tempo, di produrre nuovi rallentamenti dei processi. Partirò anch'io dall'abuso d'ufficio, vero punto critico di questo provvedimento. «Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona o entità»: così recita l'articolo 19 della Convenzione di Merida, caposaldo per la lotta alla corruzione; una convenzione adottata nel 2003 e ratificata nel nostro Paese nel 2009. Inutile girarci intorno: il disegno di legge che oggi ci proponete è in aperto contrasto con questa Convenzione, così come con i suoi principi e le sue disposizioni. Cancellare la fattispecie d'abuso d'ufficio - come ha ricordato nelle audizioni alla Camera il procuratore nazionale antimafia Melillo, ma anche nelle Commissioni - esporrebbe l'Italia al rischio di apparire fonte di indebolimento del sistema di incriminazione, proprio mentre il Paese si appresta a utilizzare ingenti risorse, quelle del PNNR, che sono anche il frutto di tasse pagate da cittadini di altri Stati europei *(Applausi)*, oltre che dai cittadini italiani. Anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione di questo Paese, Giuseppe Busia, ha sottolineato il *vulnus* normativo che rischia di generarsi con questa modifica normativa.

L'Autorità anticorruzione di questo Paese ha anche ricordato come i contenuti di questo disegno di legge mettono il nostro Paese in una posizione ambigua, a rischio di incoerenza rispetto all'ordinamento internazionale. Busia ci dice: «Con un decreto legislativo dell'ottobre 2022, abbiamo giustificato il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite e della direttiva europea sulla protezione interessi finanziari, in materia di peculato, inserendo un rinvio all'abuso d'ufficio, che verrebbe meno nel caso di abrogazione». Aggiungo che dobbiamo ricordare in quest'Aula che le norme sull'abuso d'ufficio hanno già subìto una modifica - lo hanno detto meglio di me i colleghi che mi hanno preceduto - per andare incontro alla cosiddetta paura della firma, tanto che già oggi le norme circoscrivono il campo della rilevanza penale a condotte prive di qualsiasi discrezionalità, e questo lo sappiamo bene; un discorso che si può analogamente fare per il traffico illecito di influenze, una norma recentissima che questa maggioranza ha sentito il dovere incomprensibile di modificare. Le modifiche del reato di abuso d'ufficio, introdotte nel 2020, avevano già raccolto osservazioni arrivate dai sindaci e dal mondo della pubblica amministrazione. Va anche segnalato il lavoro emendativo che il Gruppo Partito Democratico ha condotto in Commissione giustizia per scongiurare un'abolizione totale del reato di abuso d'ufficio; un lavoro di proposta che, però, si è scontrato con il muro alzato dalla maggioranza e dal ministro Nordio, sordo alle richieste di mantenere il nostro Paese al passo con gli Stati europei, evitando l'abrogazione di una norma che avrà inevitabili ricadute negative sulla tenuta dell'etica pubblica e sulla tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini. Allo stesso modo, non si comprende la scelta di togliere rilevanza penale alla condotta di millantato credito: si tratta di comportamenti certamente volti a inficiare la credibilità e l'immagine della pubblica amministrazione. I dubbi interpretativi sui margini applicativi della fattispecie, semmai, avrebbero dovuto suggerire una riscrittura, non la totale abolizione. L'analisi del disegno di legge Nordio passa anche dalla stretta che questo Governo ha voluto inserire sulle intercettazioni. Vengo al punto: con le modifiche che proponete non sarà più possibile trascrivere l'intercettazione di terze persone coinvolte nell'indagine, scelta adottata proprio per evitare che possano essere pubblicate. Da una parte, dunque, si cancellano i reati come abuso di potenza e il traffico di influenze e, dall'altro, si agisce sulla libertà di stampa. È chiaro quindi il vostro intento: da una parte, impedite che le prove entrino dentro i dibattimenti, vietando la trascrizione delle intercettazioni, e allo stesso tempo impedite che siano rese pubbliche. In questo modo, nascondendovi dietro il tentativo di impedire che vengano costruite gogne mediatiche, state impedendo che sia garantita piena trasparenza e libertà di informazione: un vero e proprio bavaglio - non ci sono altre parole per definirlo - aggravato dall'obbligo che introducete di distruggere del tutto le intercettazioni tra l'avvocato e il suo assistito, che fino ad oggi non si potevano usare nel processo, né tantomeno pubblicare, ma comunque restavano agli atti. misure, quelle contenute nel disegno di legge oggi in discussione, che si aggiungono a quanto già prodotto fino ad oggi da questo Governo e alla parola del ministro Nordio, che ha riferito in quest'Aula non più tardi di due settimane fa. Le norme sulla prescrizione, già approvate alla Camera, mettono in discussione gli impegni presi con il PNRR, con il rischio di perdere tre miliardi di finanziamenti. Soprattutto, la relazione del ministro Nordio alle Camere ha preso la forma di un gravissimo attacco alla magistratura, con accuse di mancanza di indipendenza e proclami sulla separazione delle carriere. In questo Paese, signor Presidente e colleghi, c'è una magistratura che lavora e che ogni giorno viene minacciata dalle mafie e dalla criminalità organizzata e che dovrebbe trovare sostegno nel rispetto delle diverse funzioni e non essere attaccata. Signora Presidente, mi avvio a concludere. Dicevo all'inizio del mio intervento che con questo disegno di legge emerge non una visione riformatrice della giustizia, ma anzi una grande confusione; non si offrono risposte ai veri problemi dell'ordinamento giudiziario, dalla carenza delle risorse e di personale fino alla durata dei processi. Emerge però con drammatica chiarezza un disegno politico di questa maggioranza; un disegno che si traduce con la precisa volontà di indebolire alcuni meccanismi di controllo istituzionale e civico sulla gestione del potere pubblico. Non si può dire in altro modo: si va dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio e di altre norme fondamentali fino al bavaglio sulle intercettazioni. Abbiamo davanti il rischio concreto di togliere strumenti allo Stato e alla magistratura nel contrasto alla corruzione e le conseguenze, in questo caso, superano il perimetro di applicazione della giustizia e sfociano sul piano dell'etica pubblica, con il rischio che una pratica indisturbata, impunita e profittevole di svariate forme di abusi di potere, trovi ancora più spazio nel nostro Paese. È compito del legislatore garantire e curare il bene comune giustizia. I cittadini e le cittadine ci guardano e ci chiedono di avere attenzione sui grandi temi: quello della lotta alle mafie, dalla corruzione all'evasione fiscale, al conflitto di interessi e alle carceri. Il Governo guarda invece dall'altra parte. Con questo provvedimento si indeboliscono gli strumenti preventivi e repressivi per combattere condotte corruttive.

il Parlamento approvò le tre riforme cosiddette Cartabia: quella del penale, quella del civile e poi quella ordinamentale. Ricordo le parole che l'allora sottosegretario Sisto pronunciò: finalmente eravamo a un ritorno alla Costituzione; finalmente dopo tanti anni, si poteva davvero parlare di una giustizia che si colloca nel solco dei principi costituzionali. Ecco, queste erano le parole. Poi si insedia questo Governo che non ritiene di applicare quelle riforme che - come abbiamo detto anche in altre circostanze - non rappresentavano, né rappresentano certamente le migliori riforme possibili, ma ebbero un grandissimo pregio che voi, con la vostra esperienza di Governo, completamente capovolgendo. Il pregio era che per la prima volta, dopo trent'anni di guerra tra politica e magistratura, con grandi responsabilità innanzitutto della politica, a partire da quella che si riconosceva in Silvio Berlusconi

avevano approvato delle riforme di sistema; non riforme contro qualcuno o a favore di qualcuno, ma riforme - come si dice - di struttura, in grado cioè di provare ad aggredire i nodi di una giustizia ingiusta, soprattutto delle cui lacune e mancanze a pagare il prezzo sono i cittadini. Bene, che cosa avrebbe dovuto fare un Governo serio, coerente e davvero attento attento agli interessi dei cittadini e di una giustizia giusta? Secondo noi, avrebbe dovuto applicare quelle riforme, magari vederne i limiti anche sul campo, nel momento in cui venivano applicate, e magari proporre dei tagliandi al Parlamento, ma applicarle,

stabilizzare i ragazzi degli uffici del processo, perché, se non vi sbrigate a farlo - come abbiamo chiesto - fuggiranno tutti perché le proroghe sono segno di precarietà. Evidentemente, siccome hanno lavorato e hanno dato un contributo importante, la stabilizzazione è quello che può consentire

cambiato rotta e capovolto quell'impostazione, ma c'è un motivo politico per il quale lo avete fatto. Lo hanno detto molto bene, nei loro interventi, Alfredo Bazoli, Enza Rando e prima, nell'intervento sulla questione pregiudiziale, la presidente Rossomando. Vedete, c'è uno scambio

c'è qui il ministro Calderoli, che lo sa meglio di noi - se non una lesione dei poteri del Parlamento e dei poteri e del ruolo del Presidente della Repubblica? Questa riforma della giustizia che altro è, se non la lesione di alcuni principi costituzionali?

penso perché non riformare e non tipizzare ulteriormente, ma smantellare l'abuso d'ufficio significa obiettivamente dare un messaggio che va insieme all'annuncio che lo stesso ministro Nordio ha fatto di voler mettere le mani sui reati della pubblica amministrazione. questa cosa colpisce un caposaldo dello Stato di diritto e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione ed è un colpo al contrasto alla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione, che sono tra le piaghe principali del nostro Paese. Vengono calcolati da istituti europei indipendenti in 120 miliardi l'anno i costi della corruzione in questo Paese e abolire - non tipizzare ulteriormente, semmai - l'abuso d'ufficio significa dare un segnale a chi invece non fa

per gli affidamenti diretti degli appalti; avete smantellato con il nuovo codice degli appalti i controlli e avete tolto quelli concomitanti della Corte dei conti nel PNRR; avete abbassato le soglie di controllo negli appalti dei lavori pubblici, dando

il mantra della velocità: anche noi vogliamo le opere pubbliche, un'amministrazione veloce e celere, soltanto che, senza trasparenza, la velocità rischia di essere un favore ai poteri criminali, a chi non rispetta le regole, a chi non sta correttamente sul mercato *(Applausi)* e colpisce le migliaia di imprese che invece il proprio dovere lo fanno, si rimboccano le maniche, non truccano e non vogliono truccare gli appalti e non sono né concussori, né vogliono corrompere nessuno nella pubblica amministrazione. quindi una lesione di principi costituzionali, perché si inseriscono anche in altri provvedimenti. È stata ricordata da Enza Rando prima anche la stretta sulle intercettazioni: come ricordava qualche magistrato qualche giorno fa in interviste pubbliche, l'intercettazione, tra l'altro, oltre a essere un grandissimo ed efficacissimo strumento di indagine, che semmai va rafforzato e non indebolito, oltretutto oltretutto ha portato alla scoperta di reati e quindi all'adozione di misure di prevenzione, di sequestri cautelari e di confische per centinaia di miliardi, per un costo che arriva a un miliardo o poco più. anche un vantaggio per le casse dello Stato, oltre ad uno etico e morale, che è quello di combattere l'illegalità diffusa nel nostro Paese. Come

avvocati, professori universitari, insomma personalità dello Stato, alcune delle quali rischiano anche la vita nel fare il proprio dovere. Perché non li ascoltate, se vi dicono di non abolire l'abuso d'ufficio? Anche noi vogliamo difendere gli amministratori perbene, che sono la stragrande maggioranza, ma vogliamo farlo, come abbiamo fatto, con le nostre proposte di legge, cercando di togliere loro i reati omissivi impropri, le responsabilità dirette quando non sono in capo a loro, togliendo le responsabilità erariali, tutelandoli in questo senso, evitando per certi tipi di reati la sospensione immediata in caso di condanna prima dell'appello (per certi tipi di reati, non quelli di grave allarme sociale, come quelli mafiosi o di corruzione). Così si tutelano gli amministratori perbene. insieme certamente agli amministratori perbene, vogliamo tutelare i tanti cittadini perbene *(Applausi)*, ma voi questa categoria la mettete nell'ultimo angolo. Insomma, signora Presidente, c'è un disegno coerente di attacco alla Costituzione, perché si smantellano baluardi e caposaldi di lotta alla corruzione e alle mafie e al tempo stesso si cerca di dare un colpo alla separazione dei poteri, all'indipendenza della magistratura; ebbene, in questo attacco a impalcature costituzionali non poteva mancare l'attacco al contropotere per eccellenza, che è quello tutelato dall'articolo

a trasmissioni del giornalismo di inchiesta come «Report» e a importanti scrittori anticamorra come Roberto Saviano. Cosa sono questi, se non messaggi di voler mettere la mordacchia alla libera informazione?

speriamo venga mantenuta su princìpi liberali e democratici. L'Europa ci chiede di combattere la corruzione, di garantire la libertà di informazione e non di mettere in fondo alle vostre iniziative la lotta alla corruzione, la lotta alle mafie e l'attacco e la lotta per la libertà dell'informazione.

colleghi, Governo, eccoci qui di fronte ad una riforma che entrerà certamente a pieno titolo nei manuali delle università, che segnerà il percorso di tanti giuristi in erba e che sarà oggetto di molteplici commentari che ne tesseranno l'elogio. Ovviamente il mio è sarcasmo, perché non sarà così. La non riforma della giustizia targata Nordio altro non è che il paravento necessario al fine di addivenire alla depenalizzazione dell'abuso d'ufficio. Finalmente ci siete riusciti. Tutto questo inutile ginepraio di norme, questi irragionevoli meccanismi volti, da un lato, a ingolfare la macchina giudiziaria e, dall'altro, a tutelare i colletti bianchi, servono solo a mascherare quello che è il vero motivo della non riforma: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Visto che c'eravate, perché non depotenziare - ma direi anche annullare - il traffico di influenze (delitto, quest'ultimo, introdotto dal cosiddetto spazzacorrotti per rispondere a una procedura di infrazione)? Proprio nel momento in cui si accende il dibattito nell'opinione pubblica sulla necessità di giungere a meccanismi più efficaci nella lotta alla corruzione, all'aggiornamento delle disposizioni per combattere il conflitto d'interesse e alla regolamentazione delle *lobby*, voi che fate? Assolutamente l'opposto. Nel momento in cui dall'Europa ci giunge una proposta di direttiva anticorruzione, voi come rispondete? Abrogando l'abuso d'ufficio e depotenziando il traffico di influenze. Mi sembra logico, tutto molto chiaro. C'era però da immaginarselo, vista la situazione in cui versa questo Governo. È trascorso poco più di un anno dall'inizio della legislatura e non c'è un giorno, dico uno, in cui la rassegna stampa non ci restituisca fatti di estrema gravità: la ministra Santanchè sotto indagine per la gestione del gruppo Visibilia; il sottosegretario alla giustizia Delmastro rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito;

Pozzolo (una questione, tra l'altro, da chiarire in sede processuale, visti gli ultimi allarmanti sviluppi: una festicciola con un Sottosegretario, un deputato, un sindaco e non si sa quanta Polizia penitenziaria e, a distanza di tre mesi, non si riesce a conoscere la verità). tace sulle questioni aperte in Giunta, che da organo paragiurisdizionale si sta trasformando in organo politico per eccellenza, che prende decisioni salvaguardando più questioni politiche che altro. Potrebbe mai questo Governo attuare una compiuta riforma della giustizia scevra da qualsiasi tipo di condizionamento interno? Come può la maggioranza mantenere la lucidità su un tema che va a toccare la carne viva dei comportamenti dei suoi partiti? Poi arrivate voi, quelli che non sanno quello che fanno o lo sanno fin troppo bene, perché avete un disegno ben preciso e cancellate tutto.

tanto è stato detto e tanto diranno ancora i miei colleghi in seguito, ma una domanda me la pongo e l'avrei voluta porre al ministro Nordio, qualora si fosse degnato di prendere parte ed ascoltare il dibattito dell'Assemblea di oggi.

Voglio sapere se un delinquente riesce a parlare con un ministro o di un ministro o con un sindaco o di un sindaco: voglio sapere perché ci riesce e voglio altresì sapere di cosa hanno parlato. Sarà poi il giudice a stabilire se c'è un reato. Io ho però il diritto, in in quanto cittadino, di essere informato della cosa. Io voglio sapere se un Verdini qualunque pensa di poter manovrare l'Anas a suo piacimento e stare tranquillo perché si sente sicuro e protetto da suoi contatti politici *(Applausi)*, come dicevo prima, indipendentemente dagli esiti dell'inchiesta e dando per scontata e certa, nel caso specifico, la totale estraneità del ministro Salvini, per esempio. Non venite a raccontarci poi che la tutela del terzo estraneo è fatta per proteggere i cittadini comuni dall'essere sbattuti in prima pagina, perché dovreste portarci gli esempi di questi cittadini comuni sbattuti in prima pagina. Allora smettetela di considerare i cittadini degli imbecilli e smettetela di prenderli in giro. prenderli in giro. Anche questa norma tutela i colletti bianchi e imbavaglia la stampa e i giornali, al pari di quella vergognosa norma approvata poco tempo fa con cui avete deciso di impedire la pubblicazione integrale o l'estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, cosa che

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e l'annullamento del traffico di influenze oppure la regolamentazione delle *lobby* e l'aggiornamento della normativa sul conflitto di interessi, che è ferma dal 2004? Sapete quando è stata fatta la legge relativa alle incompatibilità parlamentari? Era il 1953. Non credete che sia venuto il momento di aggiornarla? È possibile che in quest'Aula siedano senatori che, invece di perseguire il mandato con disciplina ed onore, lo svolgono al fine di un proprio tornaconto tornaconto personale? La non riforma della giustizia non interviene su nessuno di questi punti. Si continua a perseguire una politica volta alla tutela dei soggetti forti piuttosto che di quelli considerati deboli. Viene totalmente dimenticato un discorso, quello dei diritti civili. Siamo riusciti a far incardinare in Commissione giustizia la questione del doppio cognome, ma vedremo come andrà a finire. Altre questioni aperte che mai verranno affrontate in questa legislatura sono la morte volontaria medicalmente assistita, la maternità surrogata solidaristica e le detenute madri. Ma non pensate che anche questi siano temi importanti per il nostro Paese? Se non fosse stato per le opposizioni, in legge di bilancio non ci sarebbe stato nulla nulla a favore delle donne. A parole, tutti bravi, ma poi, quando si tratta di andare a distribuire le risorse, è sempre meglio destinarle a microinterventi localistici, come vi abbiamo visto fare. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione e tramite lei mi rivolgo a quest'Assemblea. Negli altri Paesi questo non succede: non c'è il surreale e vergognoso dibattito che state propinando a questo Paese e reati come quelli che voi oggi decidete di cancellare ci sono e vengono perseguiti. Ma qui no: qui si si sceglie deliberatamente di correre dietro ai magistrati e non ai delinquenti *(Applausi)*, per citare un giornalista, uno dei tanti che odiate e uno dei pochi che non fa da megafono a radio Giorgia. Siete ancora in tempo per ripensarci, ma mi riesce difficile appellarmi a un vostro scatto di coscienza, per cui non lo farò. Noi abbiamo capito cosa avete in mente; i puntini li abbiamo uniti e il disegno ormai ci appare molto chiaro. Siamo e saremo qui in quest'Aula e nelle piazze, a ricordarvi che il Paese non è quello che state cercando di costruirvi su misura, a colpi di decreti e riforme

Signor Presidente, mi consenta, tramite lei, di ringraziare il ministro Calderoli per la presenza Lo voglio ringraziare perché è dovere del Governo rimanere in Aula e il ministro Calderoli è sempre rimasto in Aula, ma anche in Commissione, sui provvedimenti che riguardavano il suo Ministero: mi riferisco

non c'è il ministro Nordio in questa circostanza. Verrà domani, perché in fondo è domani che si voterà. Questa però si chiama discussione generale perché perché è lo spazio in cui tutti i parlamentari, in questo caso i senatori, possono raccontare il lavoro fatto in Commissione e le posizioni che hanno assunto, spiegare e confrontarsi, perché l'Assemblea ha una dignità.

per raccontare anche un po' di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento. Si tratta però di un rispetto, Signor Presidente, che - mi dispiace doverlo sottolineare - manca anche nei lavori in Commissione (e non per il lavoro della Presidente, che lo svolge con il ruolo istituzionale che le compete). Spesso vado nelle scuole, dove vengo invitata a raccontare il processo legislativo durante le ore dedicate alle lezioni di educazione civica (chiaramente non vado come un'esponente politica, ma come una rappresentante delle delle istituzioni). Quando sono a scuola, racconto ai ragazzi come funziona: se c'è un decreto del Governo o un disegno di legge del Governo, questo viene assegnato a una delle due Camere e poi

Chiama immediatamente gli esperti in materia, perché attua il cosiddetto percorso di audizioni: vengono cioè invitati i maggiori esperti di quella materia a dire cosa ne pensano del provvedimento che è uscito dal Governo, per portare il loro contributo e dire cosa va bene, cosa è sbagliato e dove si potrebbe migliorare. Il processo delle audizioni è fondamentale per consentire al legislatore di svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo e, sulla base delle audizioni che vengono dall'esterno

cos'è successo anche in questo caso? A fronte di tantissime posizioni degli auditi, che segnalavano una serie di errori o problematicità che questo provvedimento ha messo in evidenza, evidenza, e di un'opposizione che ha presentato una serie di emendamenti, accogliendo i suggerimenti degli esperti (quindi non partendo per partito preso, ma cercando di aiutare chirurgicamente quel provvedimento ad essere migliore), essere migliore), gli emendamenti del Partito Democratico sono stati respinti tutti al mittente e non sono stati accolti. Non sono stati accolti perché questo è un Governo che non ascolta e non si mette nella condizione di dire che l'opposizione può portare il suo contributo e la sua voce *(Applausi)*, ma pensa in partenza che l'opposizione abbia una visione pregiudizievole o pregiudiziale nei confronti del provvedimento e quindi tutto debba essere respinto. Perché dico questo? Ne ho Ne ho sentite tante anch'io. Ha fatto bene prima il collega Bazoli, nel suo lungo, appassionato e preciso intervento, a specificare. Attribuiscono al partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, posizioni che non sono vere. Per esempio, ci dicono che siamo contrari all'abolizione dell'abuso d'ufficio. Il Partito Democratico su questo ha sempre avuto una posizione chiara: ha detto dove quella norma funzionava ed era necessario che rimanesse e ha detto dove quella norma poteva rischiare di creare problemi. E l'ha detto non a parole, ma attraverso una serie di provvedimenti che ha depositato nella scorsa e anche in questa legislatura, in cui sostanzialmente abbiamo provato a intervenire puntualmente. C'è un termine che è stato utilizzato nel dibattito: è necessario che l'abuso d'ufficio sia tipizzato, cioè circoscritto e individuato per alcuni aspetti. Noi dicevamo di accogliere l'allarme dei sindaci e degli amministratori, che ci avvertivano di stare attenti rispetto a questa questione, poi però vi è tutto il resto del mondo. Il primo interesse di chi legifera dovrebbe essere quello di mettere al centro i cittadini. allora questa domanda all'esponente del Governo, sempre tramite lei, signor Presidente: con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, in questo modo, i cittadini sono più o meno tutelati?

*(Applausi)*. Il collega Bazoli, che è Capogruppo in Commissione giustizia, prima ha elencato chi può commettere un abuso d'ufficio. È vero, possono essere i sindaci, ma l'abuso d'ufficio è commesso da chi svolge un incarico dirigenziale in qualsiasi ambito della pubblica amministrazione

O pensiamo che tutti quei fatti per cui i cittadini avevano bisogno di una copertura verranno eliminati automaticamente, che non vi sarà più nessun problema e che quindi i cittadini staranno tutti bene? bene? Il legislatore svolge bene il suo lavoro se si prende cura ed ha a cuore anche questa posizione. Mi spiace, ma con questo provvedimento il ministro Nordio non fa del bene ai cittadini. il ministro Nordio e questo Governo avrebbero dovuto accogliere la proposta che ha fatto il Partito Democratico, salvaguardando i sindaci e i nostri

la porta di un asilo nido non aveva funzionato bene e un bambino era rimasto con il dito incastrato. Questa cosa è una responsabilità della sindaca? Chi può dire che sia stata una responsabilità della sindaca? Nessuno qui dentro lo vuole dire e il Partito Democratico, proprio per evitare che si possano verificare ancora situazioni di questa natura, è intervenuto con una proposta per evitare davvero che un atto del genere potesse essere attribuito a un amministratore o a un'amministratrice. Questo significa andare incontro ai nostri amministratori, aiutarli, sostenerli e dare loro una mano, senza eliminare tutto ciò che può servire ai cittadini per far sentire la loro voce. Questo però è un problema che la maggioranza ha, perché è molto più semplice fare norme populiste, che si comunicano immediatamente, piuttosto che intervenire direttamente su argomenti e norme di legge che magari non funzionano completamente. Questo però non interessa, signor Presidente. sono anche un po' pignola di carattere e, sempre pensando a come pormi nei confronti di questo provvedimento del ministro Nordio,

abbiamo lavorato a tutta una serie di grandi riforme che hanno toccato gli ambiti della giustizia. Avendo fatto tutti quei cambiamenti,

Allora, nella mia pignoleria, sono andata a vedere se ci fossero dati relativi al frutto delle riforme che erano state fatte nella scorsa legislatura li ho trovati, Presidente, perché sono diffusi dal Ministero della giustizia e c'è una bellissima tabella. Le statistiche sono chiare e ci dicono che, ad esempio, rispetto al problema numero uno della giustizia italiana, cioè l'efficienza e la durata processi, le riforme fatte nella scorsa legislatura stanno producendo effetti veramente positivi. Secondo i dati che però mi risulta siano passati molto sottotraccia, perché quando ci sono delle belle notizie mica le si sponsorizzano o si raccontano - risulta al momento che, considerato il 2019 come punto di riferimento,

al Vice Ministro e Sottosegretario della giustizia che sono presenti in questo momento e che purtroppo si sono persi la prima parte del mio intervento, ma farò modo di consegnargliela, in modo tale che possano apprezzarne gli stimoli:

Allora perché questo Governo, anziché implementare una riforma che stava funzionando, lavorare su quei temi o occuparsi di quelli e dei problemi della giustizia, sta nuovamente sventolando una bandierina di propaganda che serve, perché

a una riforma con norme così discusse, che hanno dato vita a più di una controversia non tra le parti, opposizione e maggioranza, ma nella magistratura

che ci fosse o meno - della giustizia. Questo ha comportato che il nostro Paese non abbia legiferato sulla macchina della giustizia, sulla certezza del diritto, su un processo giusto, sulla durata dei processi, implementando il numero dei magistrati e degli operatori della

Non averlo fatto ha comportato, negli anni, una situazione di grandissimo deterioramento non solo delle nostre istituzioni, ma della nostra economia. Io sono in Commissione bilancio

di far funzionare bene la macchina della giustizia - processo civile, processo penale, certezza delle norme e certezza del diritto - il Paese non riesce Paese non riesce ad attrarre investimenti e fa fuggire il mondo dell'impresa. Quante volte abbiamo sentito dire questo in Italia? In quanti dibattiti è stato detto che uno dei temi principali della lentezza del sistema economico italiano e della sua capacità produttiva è dovuto anche a giustizia e pubblica amministrazione? Sono Sono trent'anni che sentiamo parlare di riforme della giustizia e trent'anni che sentiamo parlare di semplificazioni normative, tant'è vero che, ogni volta che c'è una legge sulla semplificazione, lo dico a titolo personale, mi spavento, perché penso sempre che entreremo in una nuova fase complicatissima, di cui gli italiani diranno che

Severino. In quel momento non fu un caso che si intervenisse sulla corruzione, sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze, in una fase di recessione dell'economia italiana, in cui si ritenne che intervenire in quest'ambito fosse una

Abbiamo poi tutta la stagione dell'istituzione delle agenzie, tra le quali l'Anticorruzione. Le norme anticorruzione hanno attraversato i Ministeri e sono diventate, dopo dieci anni, di uso comune nella pratica amministrativa, il che non era semplice. Poi arriviamo all'altro momento eccezionale della vita italiana, di un altro Governo di emergenza nazionale, quello del presidente Draghi, nel quale erano presenti tutte le parti politiche eccetto una, quella del Presidente del Consiglio, con le leggi Cartabia, che - guardate - andavano ossessivamente nell'indirizzo di mettere i punti che ci servivano

Ora, come la collega Malpezzi (siamo due precisine), anch'io ho preso il resoconto del Ministero della giustizia

positivi che ci sono stati dopo la legge Cartabia nel raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si era data, mi sarei aspettata dal ministro Nordio - che tra l'altro tutti conosciamo come persona ragionevole

c'è un *vulnus* che è quello del personale. C'è la necessità di un rafforzamento del personale attraverso assunzioni, concorsi, velocizzazione delle procedure di assunzione, stanziamento di fondi *ad hoc* nella legge di bilancio - questa questa sconosciuta - per far raggiungere questi obiettivi di efficienza che - ricordiamolo - avrebbero una ricaduta nel nostro Paese come effetto leva di diversi miliardi. E non parliamo ancora della lotta alla corruzione, ma stiamo parlando semplicemente di quanto l'efficienza del sistema amministrativo e del sistema processuale impatti sull'economia. quindi, aspettati questo. Sinceramente, essendo sempre stata una tifosa del sistema accusatorio, mi sarei anche aspettata - e spero che arrivi - una proposta di riforma

Alla fine questa riforma tanto sbandierata che roba è? È l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, di cui è stato detto moltissimo e qualcos'altro dirò. È l'eliminazione del traffico di influenze, l'ennesimo rimaneggiamento della prescrizione, come se quattro riforme in sette anni non fossero più che sufficienti. Sfido chiunque

di ristampe. C'è poi il tema delle intercettazioni, che è uno di quei temi che vanno sempre di moda. E queste sono le grandi riforme?

a tutto tondo, che ha preso i voti degli italiani - dopo un anno e quattro mesi si sarebbe aspettato un progetto di riforma autenticamente rivoluzionario e non una cosetta così, che è più di bandiera che altro.

che una parte o l'altra si possa offendere per qualcosa che le piace o non è nel proprio piccolo e personale programma elettorale,

la vedremo? Ad oggi non abbiamo neanche una bozza, eppure di bozze ne girano tantissime. Abbiamo tolto qualcosa e non abbiamo messo niente, con l'idea di fissare una bandierina. Attenzione: quando si

vecchissime, anacronistiche, che oggi non hanno più senso né tra la gente né tra gli operatori. Presidente, da giurista non riesco davvero a nascondere una sensazione di sconcerto di fronte a questa riforma della giustizia che sta ancora una volta dimostrando

Capita, quindi, che troviamo un Governo giustizialista e manettaro quando si deve fare un provvedimento sui ragazzi dei *rave party*; un Governo che vuole usare la logica del manganello e della repressione quando si tratta di provvedere sui ragazzi delle periferie e mi sto riferendo ovviamente al decreto-legge Caivano. Però, poi, all'improvviso, lo stesso Governo viene preso da una sorta di timore reverenziale quando si tratta di lottare contro le grandi organizzazioni criminali o di combattere la corruzione. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto anche quando vi siete occupati dell'ergastolo ostativo: avete fatto un regalo alle grandi associazioni per delinquere che sono finalizzate a commettere reati come quelli della corruzione. Adesso siamo arrivati anche a una perla giuridica. Voi dovete creare legalità e lo fate con la cancellazione del reato dell'abuso d'ufficio: siete arrivati alla *abolitio criminis* come una soluzione ai problemi. ai problemi. Il problema del reato di abuso d'ufficio era che ci sono troppe assoluzioni e poche condanne? Allora cosa decidete di punire: soltanto quello che le statistiche vi dicono che può continuare a essere perseguito, o è il disvalore sociale della condotta che volete punire? Dentro a questo nome rassicurante - riforma della giustizia - i cittadini si aspettano qualcosa di innovativo, qualcosa che vuole finalmente mettere fine ai problemi dei cittadini. Prima di me ha parlato la collega Bevilacqua, che vi vi rendete conto di cosa vogliono i cittadini quando dite che la riforma della giustizia è da essi attesa. I cittadini vogliono una riforma della giustizia che faccia funzionare i processi; vogliono sapere che la giustizia civile possa concludere un processo in tempi ragionevoli; vogliono che la giustizia si occupi di combattere la corruzione e la criminalità

In passato volevate anche cancellare i processi. Vi ricordate la prescrizione breve? Ecco, questa è la modalità che sta adottando questo Governo. Così facendo, non si tutelano le vittime. Ricordo male io male io o in Commissione sembravamo tutti d'accordo nel voler inserire nella nostra Costituzione la tutela delle vittime danneggiate dal reato e delle persone che sono state offese dal reato? Lo ricordo io o eravamo tutti d'accordo? Oppure avete cambiato idea? Guardate che scrivere questo principio nella Costituzione non è una questione di *drafting*: significa far diventare uno dei valori fondanti del nostro Paese, uno dei valori dell'Italia, la tutela della vittima dei reati, mentre qui voi vi state solo ed esclusivamente preoccupando di una visione garantisca che tutela soltanto chi può aver commesso dei reati. Si sta confondendo il concetto di impunità con il concetto di responsabilità. Si ha paura del processo, si ha paura del sistema giudiziario che invece è un sistema che è vicino ai cittadini. Io credo che oggi questa maggioranza sia di fronte a un bivio. Può decidere di cambiare strada. Ciò significa ascoltare quello che dicono i cittadini, perché i cittadini i cittadini vogliono una riforma della giustizia. Non vogliono questa riforma della giustizia, ma vogliono una riforma della giustizia efficiente. Vi siete accorti che le imprese non investono più in Italia? Se esse non investono più in Italia, i problemi sono sempre gli stessi. Sì, certo, abbiamo il problema delle infrastrutture sulle quali non avete voluto fare nulla quando avete approvato l'autonomia differenziata. Ma c'è anche il problema della giustizia che non funziona e, se abbiamo un sistema giudiziario cronicamente nell'emergenza, La linea che avete preso è però quella del depotenziamento. Voi state togliendo le armi alle procure per poter combattere la criminalità.

fa parte dello Stato di diritto. Quando però il garantismo travalica il buon senso e sconfina in qualcosa che rasenta l'assurdo, allora non è più un principio di legalità: diventa la perversione della legalità.

la bilancia è simbolo dell'equilibrio. L'ago della bilancia non può essere spostato né verso il garantismo né verso il giustizialismo. L'ago della bilancia deve essere in equilibrio: dobbiamo trovare un modo per cui lo Stato deve evitare che siano condannate persone innocenti, ma deve assicurare alla giustizia i delinquenti e garantire la tutela dei diritti delle vittime dei reati. Un Paese in cui non funziona la giustizia è destinato al declino e noi, come MoVimento 5 Stelle, ci stiamo battendo da tempo. Vi ricorderete che nella scorsa legislatura io ero in Commissione giustizia e che noi ci siamo battuti per la cosiddetta spazza corrotti. Voi vi siete messi di traverso, perché vi dava fastidio fare delle leggi che avrebbero messo in ginocchio quel sistema di corruzione che ci caratterizza. Sono stato a Bruxelles qualche settimana fa. L'Europa ci ha riconosciuto di aver fatto passi avanti nella lotta alla corruzione e ci ha anche detto che questo ancora non basta. Quei passi avanti li abbiamo fatti grazie al MoVimento 5 Stelle che ha approvato la legge spazza corrotti. So bene che non cambierete idea. Ma, qualunque sia la vostra decisione di oggi, vi pregherei di non diffondere tra la popolazione l'idea che il sistema giudiziario sia l'unico nemico da combattere, perché i nemici da combattere non sono quelli che ci fate vedere voi, non sono gli immigrati, non sono i ragazzi dei *rave party*. I nemici da combattere sono quelli che voi non avete ancora avuto mai il coraggio di combattere seriamente.

come risulta evidente anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, oggi discutiamo di un provvedimento che, nell'affrontare una serie di questioni reali, non fa altro che alimentare nuove distorsioni nel funzionamento della giustizia. Da tempo i sindaci chiedono non semplicemente l'eliminazione del reato dell'abuso d'ufficio, ma la definizione di un perimetro certo. Anche perché quando il 93 per cento delle inchieste non arriva neanche a giudizio, è doveroso sollevare dubbi sul reato nell'equilibrio dell'ordinamento giuridico; reato che invece esiste nelle conseguenze, prima tra tutte la paura di agire, ovverosia il dilemma quotidiano di sindaci e dirigenti che devono decidere se firmare un atto rischiando l'abuso d'ufficio o non firmarlo, rischiando l'omissione in atti d'ufficio. Ricordo che la prima riforma del reato risale al 1990, anno in cui il reato era stato specificato rispetto a una precedente formulazione generica che puniva il pubblico ufficiale che causava un danno o un vantaggio ad altre persone abusando dei propri poteri. Poi è cambiato nuovamente nel 1997, quando venne eliminata la distinzione tra vantaggio patrimoniale e non patrimoniale; ed è stato modificato di nuovo nel 2020, con l'ulteriore precisazione che l'abuso d'ufficio si realizza solo se si violano specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità. Il testo vigente chiede, tra le tante cose, la doppia ingiustizia, ovvero la condotta deve essere contraria alla legge, ma anche l'evento deve essere contrario all'ordinamento. Oggi voi scegliete la strada della cancellazione; una strada demagogica che viene contraddetta nei fatti, ad esempio dalle recenti richieste di sottoscrizione di gravosi impegni, assunzioni di responsabilità antifrode e altro, da parte dei sindaci sui progetti del PNRR. La cancellazione non risolve la questione sia dal lato della tutela degli amministratori sia rispetto al contrasto alla corruzione. Per i sindaci i problemi sono legati al sistema generale delle responsabilità e il nodo il nodo principale riguarda il TUEL per evitare che i sindaci rispondano di tutto quello che accade. Faccio l'esempio di ciò che è accaduto due anni fa alla sindaca di Crema - lo ricordava prima la senatrice Malpezzi - che ricevette un avviso di garanzia perché un bambino dell'asilo si era ferito mettendo le dita nel cardine della porta tagliafuoco. Analogamente, bisogna rivedere alcune norme della cosiddetta legge Severino ed escludere la responsabilità erariale dei primi cittadini, se non per dolo. Sono tutti aspetti che, come Partito Democratico, avevamo sottoposto con una serie di emendamenti, che sono stati respinti. La cancellazione *tout court* del reato rischia di ingenerare un vuoto in un Paese che è appena quarantunesimo nel mondo nella classifica della corruzione, con il rischio di presentarsi anche a livello internazionale con grande imbarazzo per il contrasto con la Convenzione di Merida e in violazione delle direttive europee, come ha ben spiegato il senatore Bazoli. Anche sulla pubblicazione delle intercettazioni, la sensazione è quella di assistere a un dibattito vecchio e strumentale che in gran parte è stato superato con la cosiddetta riforma Orlando del 2017. Con quella riforma, assieme alla successiva del Governo Conte II, si è riusciti a costruire un meccanismo che ha evitato quantomeno gli abusi più gravi, e questo grazie alla creazione di un archivio riservato nel quale vengono custodite tutte le intercettazioni. Le parti del processo possono solo ascoltarle e non ottenere copie. Entrano nel processo solo quelle che il giudice, sentite le parti, ritiene rilevanti per l'accertamento del reato. Questo sistema va eliminando gran parte dei rischi di cui si continua a parlare. Concordiamo sulla regolamentazione molto rigorosa dei colloqui tra imputato e difensori, perché ovviamente il diritto alla difesa è sacro. Ma, d'altra parte, contestiamo il rischio che si sottragga senza limiti ai cittadini il diritto all'informazione rispetto ai comportamenti di chi ricopre incarichi pubblici. Così come contestiamo la campagna sui costi della macchina giudiziaria, che sinistramente ricorda altre campagne populiste che, nel colpire la politica, hanno colpito il funzionamento della democrazia. Con l'idea del *budget*, il potere esecutivo non solo interferisce con l'azione giudiziaria, ma dice anche che i princìpi assoluti e basilari di uno Stato moderno possono essere subordinati a condizioni di ordine economico; un messaggio che colpisce le fondamenta del patto sociale e annacqua la funzione riparatrice della giustizia agli occhi dei più deboli. Ma, se proprio si vuole accettare questo gioco dei costi delle intercettazioni, va ricordato che dalle inchieste l'Erario e i Ministeri della giustizia e dell'interno ne hanno tratto beneficio. A Napoli, ad esempio, la spesa complessiva nel 2023 per effettuare intercettazioni è di 5,89 milioni, ma il valore dei beni mobili e immobili sequestrati è di 197 milioni. A Reggio Calabria sono stati spesi 7,9 milioni, ma sono stati sequestrati e confiscati beni e contanti per 825 milioni. A Milano, su una spesa di 10 milioni, si contano sequestri per centinaia di milioni. da discutere su quante tonnellate di droga vengono intercettate e distrutte e sul relativo valore di attenuazione del danno: un parametro incalcolabile. L'altra faccia di questo populismo è la chiave penale della logica emozionale, che porta ogni conflitto o emergenza ad essere affrontati con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato o con l'inasprimento delle pene, dai *rave* al degrado delle periferie, ai migranti, alla tutela degli animali, alla gestazione per altri e così via. Ma nel frattempo il sistema giudiziario viene privato degli strumenti necessari per farvi fronte. Un caso su tutti: nelle ultime norme contro i femminicidi si è esteso l'uso del braccialetto elettronico e si sono ampliati i poteri di ammonimento del questore ed è stato introdotto il codice rosso rinforzato. Ma non un solo euro è stato destinato a tutto questo, tanto che siamo dovuti intervenire noi per metterci una pezza, destinando le risorse dell'opposizione in legge di bilancio per garantire almeno in parte queste attività. Si insegue questa logica e intanto nelle carceri: sempre più affollate, si consuma un suicidio ogni due giorni. Costruiremo nuove carceri, è la risposta del ministro Nordio, senza dire una parola sulle misure alternative alla detenzione, senza dare una speranza a chi oggi è privato della dignità. Il vostro modello di giustizia riflette una precisa concezione: una giustizia che si accanisce sui deboli, meglio se collegabili a una qualunque diversità, e che si mostra molle verso tutti gli altri, rasentando un'impunità venduta all'opinione pubblica come garantismo; una giustizia piegata ai *desiderata* di un potere esecutivo e alla sua idea di società, con buona pace della certezza del diritto, della lentezza dei processi, dei veri diritti degli imputati e anche dei condannati. Presidente, a tutto questo noi continueremo a opporci. Presidente, colleghi, noi siamo molto perplessi di fronte a questo provvedimento. Lo hanno ben detto i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti in precedenza e anche i rappresentanti di altri Gruppi di opposizione. Ci convince molto poco il fatto che l'intenzione vera che ha mosso la maggioranza nel portare avanti questa iniziativa ha a che fare con il triplice baratto che si sta organizzando all'interno della maggioranza; un triplice baratto che, come è sempre più chiaro, punta, sulla pelle dei cittadini e del Paese, anche degli equilibri istituzionali e legislativi, a dare a ciascuna anima della maggioranza una soddisfazione simbolica, una bandierina da agitare. Alla Lega si dà l'autonomia differenziata, fregandosene degli effetti che l'autonomia differenziata ha sull'unità nazionale e sulla possibilità di garantire eguali diritti sociali e civili in tutte le parti del Paese. A Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, seppure a malincuore, perché capiscono che si realizza una concentrazione eccessiva di potere nelle mani di una sola persona, danno il premierato e l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e questo per permettere ai rappresentanti di Fratelli d'Italia di sventolare, alla vigilia delle elezioni europee e anche dopo, la bandierina dell'elezione diretta di un capo. A Forza Italia, che in questo triplice baratto è il partito che esce peggio, si dà da si dà da agitare la bandierina del coronamento di una lunga battaglia, quasi ossessiva e molto ideologica, che questo partito nel corso degli anni ha condotto contro il reato di abuso d'ufficio. È evidente e tutti sono in grado di leggere le vicende politiche per quelle che sono realmente. Tutti noi comprendiamo che far funzionare una maggioranza pluripartitica non è facile e che le concessioni reciproche sono all'ordine del giorno quando esistono delle coalizioni. Ci dobbiamo, però, sempre domandare

offensivo nei confronti di nessuno. Il prezzo che il Paese paga è un prezzo alto, perché è un prezzo alto quello che comporta l'autonomia differenziata così come l'ha concepita e portata avanti il ministro Calderoli; perché è alto lo squilibrio costituzionale che si produce con il premierato. Avremo occasione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in Commissione e in Aula, di parlarne a lungo. È un prezzo alto la lesione agli equilibri del sistema del diritto penale che questo provvedimento comporta; un provvedimento che, riferendomi soprattutto all'abolizione del reato di abuso di ufficio, è allo stesso tempo - come ha detto bene il collega Bazoli - rozzo, tecnicamente grossolano, mal scritto, ideologico, pericoloso. Soprattutto, è un provvedimento che realizza allo stesso tempo un contrasto molto forte tra la legislazione italiana come sarà, se questo provvedimento diventerà

E soprattutto, si realizzano un contrasto molto forte con il contenuto di alcune convenzioni internazionali, alle quali siamo obbligati a conformarci sulla base di un articolo della nostra Costituzione, e un contrasto con una direttiva europea in corso di approvazione. Ci isoliamo anche a livello internazionale con questa iniziativa, oltre ad approvare un provvedimento completamente sbagliato, che non merita che si scomodi l'appellativo di garantista. Questa non è un'iniziativa garantista: è un'iniziativa che fa danni, che provoca un disastro nella nostra legislazione e che punta alla repressione di reati contro la pubblica amministrazione. Il cittadino viene lasciato - com'è stato ben detto anche da altri - completamente indifeso di fronte a funzionari pubblici, dipendenti della pubblica amministrazione o rappresentanti delle istituzioni che compiano degli abusi della propria posizione, cioè che facciano un uso smodato e criminale, perché illegale, del loro potere. Che senso ha tutto questo? Senza tirare in ballo - come giustamente è stato fatto - l'eterogenesi dei fini, che ci sarà. sarà. Chi oggi spazza via dal nostro ordinamento penale l'abuso d'ufficio, credendo in questo modo di cancellare le iscrizioni nel registro degli indagati di politici e funzionari che operano nelle pubbliche amministrazioni per il reato di abuso d'ufficio, in realtà creerà una situazione in cui probabilmente esploderanno le iscrizioni nel registro degli indagati per altri reati e per di più per reati di più grave entità e puniti più duramente dell'abuso d'ufficio. Quindi, ci sono anche una certa leggerezza e un modo di fare maldestro dietro a questa iniziativa e, non soltanto il carattere ideologico delle mosse che sono state compiute. Io credo che si dovesse procedere, anche di fronte ad alcune richieste accorate di intervenire sulla materia che venivano dalla comunità degli amministratori locali, in tutt'altra maniera cioè in maniera equilibrata e non dottrinaria dottrinaria e dogmatica. Cosa si poteva fare, intervenendo in maniera equilibrata? Si poteva proseguire lungo la strada che, con la riforma del 2020, ha dimostrato di dare

agire in maniera da ritagliare in modo migliore questa fattispecie di reato all'interno del codice penale, probabilmente si sarebbe potuto ottenere, con un consenso largo, un risultato importante e positivo. Invece, si è deciso di procedere a colpi di maggioranza, con la conseguenza che si otterrà probabilmente un risultato risultato molto negativo per tutto il Paese, per lo Stato di diritto e per la possibilità dei cittadini di essere difesi dagli abusi di chi esercita il potere pubblico. Credo anche che un segno - ed è l'ultima cosa che dico della maniera errata di andare avanti su questo tema che la maggioranza ha messo in campo sia l'assoluta disattenzione che è stata riservata ad alcune proposte che il Partito Democratico ha portato

sia presentando emendamenti, quando si è arrivati alla discussione specifica del provvedimento. Per esempio, la domanda che voglio rivolgere ai rappresentanti del Governo che hanno la pazienza e la cortesia di ascoltarci è in

distinguendo meglio tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, potrebbe davvero portare a un risultato che liberi gli amministratori locali dal terrore della firma e dall'effetto paralizzante di essere considerati responsabili oggettivi di qualsiasi cosa di negativo accada nel loro territorio. Non è l'abuso d'ufficio, ma è questo tipo di problemi che davvero crea difficoltà e ostacoli nell'esercizio quotidiano delle funzioni da parte degli amministratori locali. Io però non ho notizia che la riforma del TUEL vada avanti. Il tempo passa e non si fa niente e intanto si continuano a sventolare bandierine di vario genere nel più completo disinteresse degli effetti concreti di quello che si fa. Un'altra norma che noi avevamo

dei sindaci anche dopo condanne di primo grado, salvo che non si sia di fronte a fattispecie di reato molto gravi. Anche in questo caso siamo di fronte a un atteggiamento che non so nemmeno giudicare. Si è alimentata contro questa legge una tale campagna di furore ideologico che o si abbatte del tutto - e sarebbe sbagliato - o non si riesce ad ammettere che si può cambiarne un pezzo per migliorare la situazione, perché ormai la si è descritta come male assoluto e il male assoluto, per definizione, non è Siamo di fronte all'ennesimo caso di una maggioranza che resta schiava e prigioniera degli *slogan* con cui ha impostato la campagna elettorale e che una volta vinte le elezioni e andata al Governo, di quegli *slogan* non riesce più a a sbarazzarsi e a fare a meno, con effetti negativi per il Paese. Per tutte queste ragioni la nostra opinione su questo provvedimento è estremamente negativa. Crediamo che non si stia rendendo un buon servizio al nostro Paese. Non aumenterà l'efficienza della pubblica amministrazione, ma aumenteranno solo

ideato dal Governo Meloni. È una riforma che non guarda ai reali problemi sentiti dai cittadini italiani, che riguardano la durata dei processi, le condizioni delle carceri, la riabilitazione e il reinserimento, dopo aver scontato una pena, all'interno del tessuto sociale. No, di tutto questo non ci occupiamo mai. Invece ci occupiamo di un tassello che chiarisce ancora, come se ce ne fosse bisogno, che il disegno del Governo sia creare una giustizia debole con i forti e forte con i deboli, volta ad indebolire l'indipendenza della magistratura. Mi sembra chiaro e lo vediamo nella vostra volontà di separare le carriere, cosa che nei fatti sarebbe anche inutile visto che in parte è già stato fatto con la riforma Cartabia

argomento tornerò, così come sulla stesura delle pagelle che penalizzano di sicuro i magistrati scomodi, com'era un tempo quel Giovanni Falcone del cui nome vi riempite la bocca ogni 23 maggio, ma che si rivolterebbe nella tomba se potesse vedere come state riducendo la nostra giustizia.

me. Parliamo piuttosto di intercettazioni, per esempio. Gli stessi magistrati che sono venuti in audizione le hanno definite lo strumento più efficace e importante di cui dispongono per le indagini, anche e soprattutto riguardo i reati contro la pubblica amministrazione o finanziari e fiscali. Dal 2020 ad oggi c'è già stata una riforma che mette al riparo dagli abusi delle intercettazioni. Infatti, da quella data fino ad oggi gli abusi riscontrati sono pari a zero, e lo sottolineo. Il Governo continua invece a giustificare gli interventi anche con la volontà di ridurre l'applicabilità delle intercettazioni sulla base dell'assunto che il loro utilizzo sia eccessivo e sproporzionato nel numero e nei e nei costi - parliamo addirittura dei costi - rispetto ai risultati. Sul punto c'è però da constatare che ogni anno per le intercettazioni spendiamo addirittura 200 milioni, che potrebbero sembrare sicuramente tanti, ma che andrebbero rapportati al ritorno nelle tasche dello Stato con sequestri e confische conseguenti ai reati accertati per mezzo delle intercettazioni stesse. Si chiama analisi costi-benefici, ma

grazie a confische e sequestri è stato pari a 197,9 milioni, direi un moltiplicatore esorbitante tant'è che, a quanto pare, le sole confische di Napoli vanno quasi a bilanciare il costo di tutta Italia, ma non basta. A Reggio Calabria, sono stati spesi 7,9 milioni a fronte di 825 825 milioni di euro in beni e contanti confiscati. A Palermo, 30,47 milioni spesi - credo tutti ben spesi - sono stati 322 i milioni di attivo, un moltiplicatore superiore a dieci, quindi la bilancia mi sembra piuttosto in attivo. però che questa maggioranza, celandosi dietro la questione dei costi, che non rappresenta un problema, starebbe nascondendo invece una preoccupazione più grave, ovvero che le intercettazioni portino ad acquisire informazioni o notizie nei confronti di persone estranee al reato e che possano in un certo qual modo riguardare personaggi di spicco dell'opinione pubblica (purtroppo a volte capita). Questa è la *ratio* sottesa ai numerosi interventi che impediscono l'utilizzazione delle intercettazioni a strascico nei confronti dei soggetti colpiti indirettamente e anche la questione del tetto di spesa delle singole procure

Rimaniamo però sulla questione dei costi e parliamo, per esempio, della legge di bilancio: cosa avete fatto in legge di bilancio per efficientare la giustizia? giustizia? Assolutamente niente. Le assunzioni che ci sono negli uffici giudiziari sono ancora quelle previste dal piano assunzioni del ministro Bonafede, che aveva previsto 15.000 unità, che stanno entrando ancora adesso in servizio, e 20.000 a tempo determinato con i fondi del PNNR, che vi piacciono tanto, ma che vi ricordo ancora una volta sono arrivati in Italia grazie al presidente Giuseppe Conte, non grazie a voi. le uniche proposte sensate negli emendamenti presentati alla legge di bilancio erano quelle del MoVimento 5 Stelle sulle assunzioni di magistrati, di personale, per mediatori culturali e funzionari

ma noi la riabilitazione e la funzione rieducativa della pena come le vogliamo mettere in atto, se gli educatori nelle carceri non li mandiamo? È evidente che per le vere esigenze non c'è spazio, ma per una norma che prevede - udite, udite - di avvertire cinque giorni prima i destinatari di misure di custodia cautelare per reati di corruzione contro la pubblica amministrazione invece ce n'è; in questo modo i ricchi e potenti avranno tempo di organizzare le loro latitanze dorate in qualche bel Paese estero, magari sulle spiagge dorate della Tunisia. Non lo so, vedete voi.

anche ai fini di taluni rapidi aggiustamenti legislativi, che riconducano la giustizia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio della società e non già di evasione. Credo che a tutti tornino in mente le parole recenti di un Ministro che parlava di opposizione giudiziaria (questo suono è facile da ricordare). Leggo inoltre che, sull'ordinamento giudiziario, le modifiche più urgenti investono la responsabilità civile per colpa dei magistrati (anche questo ci suona familiare), il divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari e la normativa per l'accesso in carriera con esami psicoattitudinali preliminari.

mi suona molto familiare rispetto alle norme anti-*rave party* e contro i sovversivi terroristi ecologisti che deturpano beni culturali e che sono stati all'attenzione di provvedimenti celeri di questo Governo. riforma del Consiglio superiore della magistratura, che dev'essere responsabile verso il Parlamento, la riforma dell'ordinamento giudiziario, per stabilire criteri di selezione per merito (le pagelle vi dicono qualcosa?) e delle promozioni dei magistrati e per imporre i limiti d'età, eccetera eccetera. questo documento non è il programma con cui si presentò alle elezioni politiche Forza Italia nel 1994, nel 2001 o più recentemente, ma è il piano di

incrementare un regime nei confronti dei migranti, costruendo di fatto nuove carceri in cui persone che hanno la semplice colpa di essere migranti vengono trattate

conto al Governo, perché in particolare l'ultima tragedia poteva essere evitata. Tornando però al concetto di deterrenza, questo Governo e questa maggioranza sembrano credere molto all'idea che un giurista americano, Cass Sunstein, ha definito la funzione espressiva della legge, *expressive function of the law*, mutuata dalla tradizione di Cesare Beccaria, per la quale è sufficiente introdurre una norma affinché essa svolga un doppio ruolo: da una parte, rappresenta un orientamento culturale per la società, perché trasferisce e identifica i valori morali della libertà; dall'altra,

lunga dottrina, teorie economiche ed analisi empiriche che dimostrano che non basta la deterrenza formale e che, in effetti, il motivo per cui le persone scelgono di violare le norme, soprattutto se lo fanno ripetutamente, è molto più complesso. Se però legittimamente ritenete che la deterrenza, quindi norme più dure, possano creare nella società un segnale di funzione espressiva della norma che cambia il comportamento degli individui, siete legittimati a fare quel tipo di legge e a seguire quel tipo di approccio.

di deterrenza, quindi che state generando, attraverso la funzione espressiva della legge, un incentivo a violare ulteriormente le norme. Diciamo non sta in piedi nello stesso ragionamento giuridico un approccio che punta alla deterrenza, come quello che ha caratterizzato tutti i vostri provvedimenti fino ad oggi (nelle materie più varie, dal *rave party* ad altro), insieme all'idea di dire che, quando si elimina un reato dal nostro codice, questo non crei *underdeterrence*, come direbbero gli americani, cioè una sottostima dell'effetto deterrenza, quindi l'induzione a commettere reati. se questo è il caso, cioè se effettivamente, attraverso l'eliminazione di un reato, qualunque esso sia, si genera un fenomeno di sottostima e di sottoefficacia della deterrenza, questo significa che c'è qualcuno nel sistema giuridico che perde una tutela. Questa è la domanda fondamentale che oggi va posta. Eliminando la questione dell'abuso d'ufficio, c'è qualcuno che perde una tutela e uno strumento di attivazione e di difesa? Siccome la risposta a questa domanda è positiva, allora chi si prende l'onere di riformare una norma che per varie ragioni ritiene non soddisfacente, scritta male o da riformulare riformula, pone cioè un tema di riforma vera? Non c'è una riforma che elimina e abroga una norma e ritiene che per questo semplicemente si stia generando un elemento di efficienza del sistema, senza togliere tutele a qualcuno. caso, vi siete affannati a citare dati secondo i quali, da un certo punto di vista, visto che gran parte delle vicende giudiziarie che riguardano l'abuso d'ufficio finiscono in un nulla di fatto, con un'archiviazione, questa sarebbe la dimostrazione del fatto che la norma non serve. Ora, a parte che se applicassimo tale principio a tutte le statistiche di questo genere, dovremmo veramente tagliare gran parte del nostro codice penale e soprattutto, come società, scegliere quale sia la percentuale accettabile di archiviazioni per mantenere o no una una norma nel nostro codice penale. A parte questo, se credete nella deterrenza, significa semplicemente che ci sono casi che si attivano; probabilmente, la norma andrebbe scritta meglio, se ci sono elementi di discrezionalità e di confusione, ma quel dato di per sé non significa nulla, anzi potrebbe essere interpretato come segnale del fatto che la norma esistente è fortemente deterrente e che eliminarla in realtà genererebbe gli incentivi contrari e quindi un incremento degli abusi. Questo per ciò che riguarda il tema della deterrenza. Ce n'è poi un altro, la cosiddetta "firmite", cioè un meccanismo di selezione avversa - così direbbero gli economisti - per il quale, rispetto al rischio di trovarsi con una responsabilità, ci sarebbe un incentivo da parte di diversi decisori pubblici a non compiere determinate azioni o a ritardarle per paura di incorrere in un possibile rischio che non riescono a stimare. Questo tema può esistere ed è tipico di tutti i casi in cui c'è un problema di eccesso di responsabilità. Ci sono tanti ambiti nei quali l'eccesso di responsabilità può creare un'inibizione all'azione, però il problema è che questo stesso meccanismo e questa stessa spiegazione stanno alla base delle riforme prospettate del TUEL e di quelle che questa maggioranza sta prospettando sul magistrato contabile. Allora, delle due l'una: non si può pensare che la norma firma sia generata da un problema soprattutto di magistratura contabile e di responsabilità e, dall'altra parte, pensare che con l'eliminazione dell'abuso d'ufficio si risolva il problema della selezione avversa per i decisori pubblici. Non ci può essere un fenomeno che ha diverse cause; può accadere, ma a questo punto andrebbe fatta una riforma in quota parte e specificato in che senso un certo tipo di di normativa incida sugli incentivi o meno dei decisori pubblici a compiere o no determinate azioni od omissioni. Tutto questo manca, perché l'analisi è partita dall'idea che intanto va eliminata questa norma e poi il resto si vede. Ecco, questo non è corretto, perché non ci permette, tra le altre cose, di analizzare i problemi e di fare un'analisi comparata delle riforme che devono essere effettuate e delle efficienze che dalla norma ci si attende. La collega Malpezzi ha citato molto bene alcuni risultati importanti che sembrano attribuibili alla riforma Cartabia. Ebbene, in questo caso un buon legislatore osserva il risultato, cerca di capire quali sono gli elementi positivi e interviene modificando delle norme, ma anche individuando gli obiettivi. Il tema della "firmite" ha troppi padri e troppo potenziale di riforme per poter essere affrontato seriamente; e ancora in quest'Aula oggi non è emersa una spiegazione chiara, logica e verificabile del motivo per il quale, una volta eliminato questo reato, si risolva il problema della selezione selezione avversa del decisore pubblico. Arrivo ad un altro punto, un po' più interessante sotto il profilo filosofico, che è quello dell'inappellabilità dal lato dell'accusa nel caso di assoluzione. Questo è un punto sul quale si può discutere, perché effettivamente l'introduzione del principio del ragionevole dubbio nel nostro ordinamento somiglia molto all'impostazione che c'è in altri sistemi di *common law*, ma allo stesso tempo questa somiglianza non si può limitare a importare una norma nel nostro ordinamento, introducendo un elemento asimmetrico, senza considerare la complessità dei sistemi. sistemi. Il sistema della *double jeopardy*, che si basa sul principio che non si può essere messi sotto processo per lo stesso reato, nei sistemi di diritto anglosassone nasce da una circostanza di economicità dell'azione giuridica, ma in una simmetria tra accusa e difesa che lì è impostata con un sistema completamente diverso. È una simmetria che fa sì che, però, dopo una condanna di primo grado, ci siano delle conseguenze. Allora, da questo punto di vista, la famosa sentenza che qui è stata criticata da parte della maggioranza ha posto un tema, e il tema dev'essere che non si può inserire in questo sistema un meccanismo... La invito a concludere, senatore introdurre questo sistema, ma che allora anche l'appellabilità dal lato dell'accusa dovrebbe avere un sentiero più ristretto, proprio per consentire tale simmetria. In conclusione, Presidente, questa non è una riforma. Una riforma della giustizia avrebbe bisogno intanto di essere tale e di guardare al sistema; qui ci sono piccoli interventi, che nascono più dalla memoria di piccole questioni che si vogliono mettere insieme che non dall'ambizione seria di cambiare e migliorare il nostro sistema della giustizia, che va dal processo e dall'indagine fino alle carceri, le tanto martoriate carceri, nelle quali abbiamo sempre meno

e, aggiungerei, di quel conflitto di interessi che aleggia tanto sulle Aule del Parlamento, ma da cui in realtà non si riesce a venire a capo. Di fatto si sta creando, Presidente, un sistema penale totalmente sbilanciato, a tutela dei soli soggetti considerati forti in società, quali i colletti bianchi, e a totale detrimento delle fasce deboli. D'altronde, cosa ci si poteva aspettare da un Ministro che, come primo provvedimento, presenta alle Camere un disegno di legge che istituisce l'arresto in flagranza per i partecipanti a un *rave party*? Che strana concezione delle priorità del Paese ha questa maggioranza, Presidente. Sulla giustizia ci troviamo all'anno zero e posso con certezza affermare che siamo di fronte all'ennesimo scempio. una riforma della giustizia, quella del ministro Nordio, che dal nostro canto non è condivisibile, in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono collegate ad appalti, mazzette e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione. il centrodestra cosa fa? Apre praterie di impunità e indossa i guanti bianchi con chi inquina le istituzioni. Lo diciamo non solo dal nostro canto, Presidente. Anche la Commissione europea, nella persona del rappresentante esecutivo dell'Unione europea, sottolinea come il pacchetto Nordio, tra le altre cose, depenalizzi un'importante forma di corruzione, rimarcando quale sarebbe l'impatto del disegno di legge in esame sull'efficacia della lotta alla corruzione, riferendosi alla cancellazione dell'abuso d'ufficio e ricordando che la massima priorità per la Commissione è proprio la lotta alla corruzione. malauguratamente il disegno di legge dovesse diventare legge, l'Italia diventerebbe l'unico Paese dell'Unione europea dove abusare del potere pubblico per scopi privati e personali sarà consentito. L'abuso d'ufficio, Presidente, è previsto e disciplinato in quasi tutti gli Stati membri. Solo nel caso della Bulgaria e della Danimarca certezza alcuna non abbiamo. L'Unione europea però è stata chiara e potremmo seriamente incorrere in un forte conflitto con Bruxelles già solo con l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Il Guardasigilli ha sottovalutato però la posizione europea e malinterpretato le parole dell'Unione. È convinto che l'unica cosa che ci sia stato chiesto sia semplicemente combattere la corruzione e nulla più. Il ministro Nordio avanza per di più, e con presunzione, che l'Italia ha un arsenale normativo per combattere la corruzione, considerando poi irrituale e impropria la considerazione della volontà dell'Unione. Al Governo italiano non è affatto chiaro che l'Europa continuerà con attenzione estrema a seguire gli sviluppi dell'*iter* legislativo del disegno di legge, del disegno di legge, che provoca imbarazzo e sconcerto anche in diversi esponenti della maggioranza. Signor Presidente, è l'ennesima occasione che dilata una spaccatura interna e propria della maggioranza, ormai presente da mesi, se non dal primo giorno della nascita di questo Governo. Come se non bastasse, il disegno di legge n. 808 prevede anche la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni, norma scritta malissimo, che crea solo insicurezza. Il numero uno dei sindacati delle toghe, il dottor Santalucia, ha criticato fortemente i provvedimenti di Nordio, attaccando il divieto di pubblicazione, anche parziale, di tutti i dialoghi che non siano stati prodotti dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzati nel corso del dibattimento e dunque anche delle conversazioni citate nelle richieste di misura cautelare del pubblico ministero. Inoltre, la parte della riforma che ha ridotto drasticamente il potere di impugnare le sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero incorre in una possibile censura di incostituzionalità. Se n'è già accennato in Aula, ma vorrei ricordare a tutti che esiste già un precedente. Era il 2006, quando la legge Pecorella, approvata dal terzo Governo Berlusconi, introdusse l'inapplicabilità delle sentenze di assoluzione di tutti i tipi di reato da parte dell'accusa, successivamente dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo. Il Governo non può non considerare l'Europa o altre posizioni autorevoli e a noi non resta che fare il possibile per fermare questo scempio, perciò ripetiamo da quasi quattro ore sempre gli stessi elementi, ma questo lo dobbiamo all'Italia onesta, signor Presidente, agli italiani onesti e alla democrazia, che meritano una giustizia autorevole e peculiare dell'uguaglianza.

ma ben altri. Come diceva il senatore Parrini, uno di questi è la ridefinizione di un perimetro certo entro il quale operare nell'ambito dello svolgimento della funzione amministrativa. *In primis*, il testo unico degli enti locali, una riforma necessaria, improcrastinabile e urgente, che delimiti con esattezza il perimetro degli organismi che sono stati eletti dai cittadini e delle funzioni degli organismi tecnici. tecnici. Troppo spesso, infatti, gli amministratori sono chiamati a surrogarsi in funzioni che non sono loro proprie. In questi giorni, mi son visto recapitare dal Ministero dell'interno una dichiarazione sostitutiva con la quale avrei dovuto attestare che, sul PNRR, nella gestione degli appalti si rispettano tutte le norme del codice, che c'è la regolarità contabile e che non si incorre in procedimenti anticorruzione. Certo che, chiedendo ad un amministratore locale di dichiarare che non terrà comportamenti illeciti come la corruzione,

precisione i compiti dei responsabili dei servizi, ai quali è attribuito un autonomo potere di spesa, di controllo e di organizzazione. Il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione non è il sindaco del Comune o il presidente della Provincia, ma, ai sensi della legge n. 190 del 2012, è colui che viene identificato dall'organo di vertice, che può essere il segretario comunale o un altro ufficio.

il profilo di applicazione dell'abuso d'ufficio, ma con norme chiare, che consentano agli amministratori di operare nell'interesse dei cittadini, nel rispetto di un testo unico degli enti locali e di tante altre norme che tutti i giorni vengono emanate o di circolari che vengono emesse dai Ministeri e rendono incerta la funzione amministrativa. Si pensi al tema che dal 1° gennaio del 2024 non esiste più lo *Smart*-CIG, una procedura agevolata per le acquisizioni da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi. La piattaforma digitale si è bloccata: per settimane i Comuni e le pubbliche amministrazioni sono stati impossibilitati ad acquistare

mattina. Gli interventi per agevolare il funzionamento della macchina amministrativa devono pertanto andare nel senso di agevolare con gli strumenti, anche amministrativi, l'espletamento di tali funzioni. Per non parlare dell'esigenza di dare alle pubbliche amministrazioni il giusto supporto in termini di personale e di risorse. Ad oggi, sentiamo tutti parlare del Patto di stabilità, ma non abbiamo ancora contezza degli effetti che avrà rispetto alla macchina amministrativa. Non ne abbiamo contezza in un momento estremamente delicato come quello attuale, in cui moltissime amministrazioni sono chiamate a dare esecuzione alle opere previste per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, progetti nati negli anni scorsi, che hanno visto una rivalutazione dei costi di esecuzione che talvolta supera anche il 30 per cento e che costringe le amministrazioni pubbliche a iniettare

all'avanzo di amministrazione, sempre che il Patto di stabilità consenta di spendere, così com'è avvenuto negli ultimi anni, parte dell'avanzo di amministrazione per la spesa per investimento. Talvolta occorre ricorrere all'indebitamento dell'ente,

rischia di implicare uno squilibrio finanziario rispetto a norme che ad oggi non sono chiare e che si rende necessario siano definite nel più breve tempo possibile. Qual è l'effetto? La responsabilità erariale da parte degli amministratori. Questo è un altro punto: chiarezza nelle disposizioni di legge e in quelle interpretative, nonché nel fatto che deve poter amministrare chiunque e non solo persone che hanno una competenza tecnica specifica, perché la funzione di sindaco la decidono gli elettori e non, a valle o a monte, le proprie competenze. È una questione di democrazia di accesso alla funzione pubblica. È questo che credo gli amministratori lamentino più di tutto, cioè quel perimetro che oggi non è definito, si continua a non voler definire e rende incerta una funzione che non è nell'interesse di chi la esercita, ma di tante donne, tanti uomini e tanti cittadini che ogni giorno hanno bisogno di beni e servizi. Concludo dicendo che ci sono interventi non che ci sono interventi non più procrastinabili che la pubblica amministrazione ritiene necessari, come la riforma e la revisione del Testo unico degli enti locali, che è un atto non più rinviabile. Sarà quello il momento in cui potremo dire che si interviene su quella che è stata definita la paura della firma, per rendere la possibilità agli amministratori di governare con la certezza delle regole, in piena trasparenza e correttezza, senza trovarsi di fronte a responsabilità che nulla hanno a che vedere con l'abuso d'ufficio.

Attualmente, il reato di abuso d'ufficio è previsto e disciplinato dall'articolo 323 del codice penale, rubricato tra i reati contro la pubblica amministrazione e, in ultima analisi, tutela l'interesse a che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio osservino determinati doveri, nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Cosa prevede esattamente questo articolo? Che sia punibile la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto. Quindi, in definitiva, il pubblico ufficiale, se rispetta la legge, non ha nulla di cui preoccuparsi: si difenderà nel processo e farà valere le proprie ragioni. Per questo il MoVimento 5 Stelle è contrario all'abrogazione di tale fattispecie di reato e concorda appieno con quanto affermato dal senatore Scarpinato nell'illustrazione della questione pregiudiziale di costituzionalità. La maggioranza, come da copione, ha necessariamente soprasseduto nell'accogliere le motivazioni di quell'atto. C'era da aspettarselo. Ciò però non sta a significare che quanto riportato nel documento non sia in un prossimo futuro accolto in altra sede. Questo rappresentava solo il primo momento di un dibattito sul punto. L'ordinamento giuridico viene in nostro soccorso e ne offre altri: il sindacato di costituzionalità del Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione e quello successivo da parte della Corte costituzionale, ferma però auspicabilmente l'ipotesi di correzione del testo alla Camera, Senza entrare nel merito della questione, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e il divieto di proporre appello da parte del pubblico ministero nei casi di assoluzione per delitto a citazione diretta potrebbero porre future questioni di compatibilità costituzionale e non solo. Sappiamo bene della proposta di direttiva UE del maggio scorso per la lotta alla corruzione che prescrive agli Stati membri la rilevanza penale dell'abuso di ufficio, in quanto reato legato a doppio filo con il microsistema corruttivo. È altrettanto noto che il reato esista nella grande maggioranza degli Stati membri. Il vuoto normativo che state andando a creare rischia quindi di prevedere successivi interventi normativi additivi, con la necessità di una riformulazione della previsione criminosa e con tutto quel che comporta in ordine al costo giuridico di questa operazione. Avremo una nuova figura di reato che varrà solo per il futuro, creando una frattura con l'abrogazione dell'articolo 123 e le relative sentenze di condanna definitiva abrogate. Insomma, il solito pasticcio all'italiana *(Applausi)* che aumenterà l'incertezza del nostro diritto e la sua affidabilità, anche considerato che le prescrizioni dell'Unione europea sulla criminalizzazione dell'abuso d'ufficio attribuiscono carattere transnazionale al reato, prevedendo la responsabilità anche per gli agenti pubblici non nazionali. Finiremo per consolidare la nostra triste nomea internazionale in tema di corruttela e favorire l'ingresso di quella internazionale che in tempi di attuazione del PNRR non è proprio il massimo. Perché non lasciare invece che producessero i loro effetti le riforme della fattispecie di reato introdotte con il decreto semplificazione del settembre 2020, che già aveva comportato una parziale *abolitio criminis*? Il nostro intervento legislativo riportava questa fattispecie criminosa entro più rigorosi criteri descrittivi, pur garantendo il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa da parte del giudice penale. L'abrogazione *tout court* del delitto in parola ha definitivamente eliminato la *ratio* per la quale il delitto era stato inserito all'interno dell'ordinamento, ovvero dare copertura penale a fatti non perseguibili sulla base di altre fattispecie. Che cosa succederà dei comportamenti che oggi risultano punibili a titolo di abuso d'ufficio? Sono fatti non privi di disvalore. Si potrebbero citare, tra le condotte affaristiche o di vantaggio, per esempio, fatti di rilascio di permessi di costruire illegittimi o di reiterata, sistematica e collusa sanatoria di abusi edilizi. È storia recente del Comune di Milano, che ha dei grossi problemi per aver allegramente consentito degli interventi edilizi non conformi. Ma, se i funzionari del Comune di Milano hanno rispettato la legge, non hanno nulla da temere. Ancora, ci sono quelli di mancata astensione, assegnazioni di posti di lavoro, incarichi di consulenza a membri della propria famiglia o a società di cui l'agente detiene partecipazioni. Ancora più preoccupanti sono i comportamenti consistenti nell'inflizione di ingiustificate offese a fondamentali diritti altrui, ancora più carichi di disvalore perché commessi da rappresentanti dello Stato, quale potrebbe essere il caso del del carabiniere che ordina a due ragazze di mostrare i loro documenti obbligandole ad attendere l'arrivo della pattuglia solo per ritorsione, perché le ragazze avevano rifiutato le sue *avance*. Ma anche per il traffico di influenze il perimetro del campo applicativo dell'incriminazione è stato notevolmente ristretto: in totale spregio delle convenzioni internazionali, il reato di traffico di influenze illecite non sarà applicabile né quando finalizzato all'abuso di ufficio in quanto abrogato, né quando finalizzato alla corruzione per l'esercizio della funzione, nonché per il conseguimento di utilità diverse da diverse da quelle patrimoniali. Proprio in un momento storico come l'attuale, ovvero quello della messa a terra del PNRR, nel quale andavano stretti i lacci contro i fenomeni corruttivi, si lasciano invece prive di copertura penale determinate condotte di così grave allarme sociale. In conclusione, date queste premesse e considerate le argomentazioni di cui alle questioni pregiudiziali proposte, nonché richiamati i contenuti delle proposte dei colleghi e del senatore Scarpinato in particolare, non posso che auspicare che la maggioranza accolga il lavoro delle opposizioni e approvi miglioramenti al testo quanto mai essenziali vista la portata del provvedimento all'esame di questa Assemblea. La speranza è l'ultima a morire. Sono un'inguaribile ottimista.

voglio aprire il mio intervento ringraziando innanzitutto tutti coloro che davvero si impegnano ogni giorno per la giustizia, per promuovere la giustizia giusta, per restituire giustizia a chi chi paga, ha pagato o ha subito il suo contrario, in testa a tutti i cittadini, quelli più inermi e poveri che poi sovraffollano le nostre carceri. Voglio ringraziare quanti governano la giustizia e fanno in modo ogni giorno, con il proprio lavoro, che possa tornare a governare le nostre vite e - come si dice - a trionfare. Voglio perciò esprimere la mia gratitudine nei confronti dei magistrati che si impegnano ogni giorno in questa direzione; nei confronti degli avvocati, spesso costretti a combattere con le inefficienze e anche con il cattivo funzionamento della giustizia. E voglio esprimere gratitudine nei confronti del personale amministrativo che incontriamo, costretto a operare in uffici fatiscenti, senza mezzi, senza strumenti a disposizione, e di chi ogni giorno entra in un carcere pensando a quanto sia cattiva e indegna la qualità della vita di chi vi è costretto e a quanto scarso sia il margine per recuperare, una volta espiata la pena, quelle persone che vi sono detenute. Il ringraziamento che garantiscono ogni giorno, anche con grandi carenze di organico, i servizi della giustizia e in particolare a chi lavora nelle carceri minorili, che abbiamo del tutto dimenticato. Il sottosegretario Ostellari, che non vedo ora qui presente, ma c'era oggi, proprio all'inizio del suo mandato aveva fatto visita al carcere minorile di Bologna e ad altri carceri minorili annunciando provvedimenti o comunque interventi che poi ancora mi sembrano non si siano visti. Oggi ho deciso di intervenire anch'io su questo enorme tema, perché penso davvero che la giustizia ci riguardi tutti, come individui e come comunità. È stato ricordato quanto sia centrale e decisivo anche per uno Stato poter garantire un sistema efficiente della giustizia e un suo governo efficace, anche nei confronti di quanti all'estero eventualmente valutano decisioni relative a grandi investimenti.

sembra che della giustizia giusta importi davvero molto poco. Lo ha dimostrato con le norme oggi sottoposte alla discussione di quest'Assemblea, che in sostanza si riassumono in una cancellazione dell'abuso d'ufficio, in una grande riduzione della portata del traffico delle influenze illecite e in un significativo ampliamento dei divieti in materia di intercettazioni, che colpirà soprattutto chi lavora nei giornali e nei quotidiani, chi in qualche modo di come vanno le cose. D'ora in poi i giornalisti potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

tra le scelte di questo Governo in materia di giustizia: davvero non si capisce bene se esiste una

stiamo addirittura discutendo dell'istituzione di un nuovo reato in relazione ai disturbi alimentari, e ciò ovviamente lascia esterrefatti pensando alla complessità del tema. D'altra parte,

sono 15 dall'inizio dell'anno, praticamente un suicidio ogni due giorni ed è stato calcolato che, se il ritmo sarà questo, purtroppo si supererà il tristissimo primato del 2022. Poco importa se Carlo Nordio, prima di diventare Ministro, aveva detto che l'errore della destra è di pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che - parole del Ministro - è criminogeno. Evidentemente questo ragionamento è valso solo per l'abuso d'ufficio.

Ecco, io penso davvero che abbiate perso una grande occasione, ma anche che il Paese stia vivendo un altro grandissimo errore. errore. Come dicevo, il sistema della giustizia meriterebbe davvero un pensiero e questo pensiero non si intravede in alcun modo dall'inizio alla fine: dall'istituzione del reato di *rave* ad oggi non si è visto un segno di luce.

nel merito del provvedimento, su cui cercherò di dire alcune cose, anche ripetendo in qualche modo gli interventi di chi mi ha preceduto e, in particolare, dei colleghi del mio Gruppo che hanno già individuato, le criticità che - a nostro avviso - sono contenute nel disegno di legge al nostro

che sia in atto una sorta di spartizione legislativa riformatrice da parte della maggioranza. Siamo partiti con il primo provvedimento, il disegno

cessione di consenso che la Lega sta avendo al Sud; a questo punto mi sembra evidente che essa torna alle proprie origini. quindi di un provvedimento di riforma che va nella direzione di una delle forze politiche di maggioranza. Anche in quel contesto però abbiamo visto che, quando abbiamo parlato di LEP, è spuntato poi un emendamento da parte di un'altra delle forze politiche di maggioranza, Fratelli d'Italia, che diventa quasi la pietra tombale sull'attuazione di quella riforma. È evidente infatti che, nel momento in cui si dice che a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei costi *standard*, prima di cedere autonomia a una Regione, si deve garantire che le risorse per tutte le altre Regioni, anche quelle che non richiedono maggiore autonomia, siano disponibili per aumentare e arrivare ai livelli essenziali delle prestazioni, significa che o sconquassiamo completamente i conti dello Stato oppure non riusciremo mai a garantire Quindi, anche all'interno del disegno riformatore della Lega, si inserisce una lotta nella maggioranza che va a bloccare quella riforma. Il secondo grande tema è la riforma costituzionale che introduce il premierato. Premesso che, nel programma di Governo del centrodestra, c'era il presidenzialismo e non il premierato, è questo un primo tradimento della della proposta elettorale del centrodestra che poi ritorna all'interno del premierato laddove il prossimo *Premier* dovrà garantire l'attuazione del programma di Governo. Governo. Sostanzialmente Giorgia Meloni non potrebbe più ripresentarsi come *Premier* perché ha già disatteso una parte del suo programma. Quello è l'elemento forte di Fratelli d'Italia che caratterizza questa azione riformatrice. vediamo oggi emendamenti presentati dal Governo e le dichiarazioni della ministra Casellati, secondo cui arriveranno altre modifiche, frutto di un equilibrio che ancora non c'è nelle forze di maggioranza, che in qualche modo bloccheranno anche quel provvedimento. Noi ce lo auguriamo, altrimenti sicuramente saranno i cittadini con il *referendum* a bloccarlo. È incredibile - e vengo quindi al disegno di legge Nordio - che,

una riforma che per noi non può contenere nulla di più lontano e distante da ciò che serve alla giustizia e della quale non salviamo sostanzialmente nulla. Citerò alcuni elementi che per noi sono molto critici e parto dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio, il punto nodale del provvedimento. Non ci sono questioni di merito che - a nostro avviso - possano essere salvate. L'abrogazione comporterà molti effetti sull'ordinamento, ma li riteniamo tutti controproducenti. Intanto l'*abolitio criminis* comporterà la cessazione degli effetti delle 3.600 sentenze di condanna già pronunciate; comporterà l'ipotetica riespansione in sede giurisprudenziale di altre fattispecie penali che, in barba ai princìpi di tassatività e certezza della pena, andranno ad assorbire per via giurisprudenziale l'*abolitio* in parola. In più, la riforma del 2020 già aveva previsto una condotta di per sé molto circostanziata, al punto da lasciare la rilevanza penale a quelle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, ossia i cittadini. La giurisprudenza della Cassazione in questi quasi quattro anni si è del resto attenuta allo spirito della riforma del 2020. Lo scarso numero di condanne è quindi prova di una capacità della giurisprudenza di selezionare rigorosamente gli abusi penalmente rilevanti e potrebbe concorrere a ridurre la paventata ansia di denuncia, oltre che a orientare le scelte dei magistrati inquirenti rafforzando la già diffusa propensione a chiedere l'archiviazione. Vi erano dunque non ragioni giuridiche per intervenire in senso abrogativo, bensì mere logiche di scambio politico. Veniamo al traffico di influenze. Il disegno di legge governativo circoscrive, svuotandone di fatto la fattispecie, la mediazione illecita unicamente all'interno della mediazione onerosa, tipizzandola sulla scorta delle sentenze della Corte di cassazione. Peccato che tali decisioni si riferiscano a una mediazione illecita finalizzata al delitto di abuso d'ufficio. Quindi, paradossalmente, da una parte si tipizza la mediazione illecita sul modello della mediazione onerosa indirizzata all'abuso d'ufficio, mentre dall'altra si abroga esplicitamente l'abuso d'ufficio. Gli effetti che questa norma produrrà sono presto detti: effetti abolitivi, con la revoca delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di cassazione per *abolitio criminis*. Ulteriori due questioni che fanno da corollario allo scempio al quale stiamo assistendo sono ravvisabili nel gip collegiale, nell'interrogatorio preventivo, oltre a quelle già citate in sede di incidente di costituzionalità. alla questione del gip collegiale, il primo pensiero sul punto riguarda i tribunali di minori dimensioni. Una siffatta introduzione comporterebbe inevitabilmente - come è già stato detto - una serie di incompatibilità a cascata e in ogni caso determinerebbe inevitabili aggravi nei tempi, nelle risorse e nei costi - in una materia, quella cautelare, ove per converso l'esigenza primaria è dare una risposta in tempi più rapidi possibili - sia nel senso di un eventuale accoglimento che di un eventuale rigetto o di applicazione di misura diversa, a maggior ragione trattandosi di decisione relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere. Tale questione andrebbe anche rapportata alle scoperture di organico della magistratura. È prevista l'assunzione di 250 gip, ma sicuramente non saranno sufficienti. Un emendamento del mio Gruppo, che elevava a 500 il numero di assunzioni, è stato incautamente bocciato. Venendo all'interrogatorio preventivo, va subito precisato che il campo di applicazione di questa nuova norma appare particolarmente ristretto, poiché la gran parte delle misure cautelari è di fatto richiesta, e proprio per la categoria dei reati per i quali viene fatta l'esclusione: reati commessi con violenza, reati in ambito di criminalità organizzata, reati codice rosso contro le fasce deboli, reati con uso di armi. In pratica, l'interrogatorio si applicherebbe unicamente ai casi in cui sussista la sola esigenza cautelare della reiterazione del reato e sarebbe escluso per una moltitudine di fattispecie violente o recanti pericoli di gravi danni materiali a persone o cose. Pertanto, quel tanto decantato effetto dirompente sulla vita delle persone verrebbe risparmiato a un numero davvero basso di cittadini. Per mezzo di tale ragionamento è possibile tracciare l'identikit dei soggetti generalmente autori del gruppo di reati ai quali è destinata la norma, ovvero i delitti commessi senza violenza, ossia tipicamente quelli dei cosiddetti colletti bianchi (reati di corruzione, illeciti finanziari e reati di bancarotta). di quelle fattispecie per le quali, non essendovi violenza, le ragioni di cautela su cui fondare l'adozione di misure coercitive vanno ricercate nella gravità dei fatti contestati, nella loro connessione a reiterazione e nella relazione diretta o indiretta con ulteriori fenomeni criminosi complessi. Un ulteriore problema dell'istituto è che, quando si avvisa un indagato della possibilità di essere afflitto da misura cautelare, il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, che in precedenza non era ravvisabile, verrebbe ad essere creato proprio in quel momento, con conseguente pregiudizio per le investigazioni e per le esigenze di tutela delle persone offese. Vista la situazione carceraria, sarebbe stato molto più saggio astenersi dal perseguire tale riforma e virare verso una compiuta riforma del sistema penitenziario. Sono quindici i morti dall'inizio dell'anno per suicidio. La soluzione - secondo la presidente Meloni - è quella di avere più posti nelle carceri e non di togliere i reati, come vuole l'opposizione; sono testuali parole della presidente Meloni. Peccato che sia proprio la maggioranza a operare al contrario: non rafforzare la presenza di carceri, ma togliere reati. In realtà, non sempre vengono tolti e qualche volta vengono aggiunti reti assurdi - la collega Zampa ne ha che poi vengono anche commentati a seconda del caso. C'è il rafforzamento del reato di blocco stradale, quando a protestare sono gli ambientalisti, e c'è il pieno supporto a chi blocca le strade quando a protestare sono altre categorie di persone. Io credo che sia evidente il quadro di spartizione delle riforme di questo Paese: a farne le spese è l'Italia. Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la sua presenza qui in Aula e per l'ascolto che ha riservato al dibattito. Diciamo la verità: noi avremmo voluto fare un dibattito vero e serio, come abbiamo fatto in altre occasioni. Il dibattito sull'autonomia differenziata è un dibattito serio e importante per il Paese; esso attiene a come declinare il principio dell'autonomia e dell'indipendenza dei territori e il loro contributo allo sviluppo del Paese. Certamente non siamo d'accordo, ma quello risulta un dibattito serio. Noi avremmo preteso che anche nel campo della giustizia il Governo avesse un'ambizione: quella di fare vere riforme e di portare avanti

subito dopo l'approvazione della legge n. 180 del 1978, il professor Basaglia noleggiò un aereo per portare i suoi pazienti, che uscivano per la prima volta dai manicomi, dai manicomi, a vedere la città dall'alto, la città che li aveva segregati, perché vedessero le cose dall'alto e avessero una visione complessiva di dove erano. a me sembra che questo provvedimento sia ancora tutto chiuso. Non vi sto dando dei matti, non voglio darvi dei matti, ma mi sembra che siate tutti chiusi dentro un recinto. L'Italia è un Paese che ha un problema enorme di corruzione, per esempio. Noi perdiamo circa il 13 per cento del PIL nei fenomeni corruttivi. L'Italia è un Paese che ha un enorme problema di giustizia, di eguaglianza dei cittadini. Una delle eredità, forse la migliore eredità della civiltà occidentale del Dopoguerra, è il costituzionalismo moderno, cioè il fatto che abbiamo costruito costituzioni importanti (quella italiana, quella tedesca, quella spagnola dopo la guerra civile), che hanno rappresentato delle direttive fondamentali per i Paesi, ai fini di uno sviluppo armonico, di uno sviluppo di uguali diritti e uguali doveri dei cittadini, di difesa delle caratteristiche dell'individuo. I miei colleghi, che sono molto più bravi e più esperti di me, in questo dibattito hanno sottolineato il fatto che questo provvedimento rischia di creare una disparità inaccettabile: un pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri e prevarica i diritti di altri cittadini rischia di rimanere impunito. È quasi certo che sarà così. Non si capisce perché, a fronte dell'enorme quantità di problemi che ha questo Paese, ci siamo concentrati sull'abuso d'ufficio. Leggo le statistiche dei dati del Ministero della giustizia. Nel 2016, erano quasi 8.000 i procedimenti per abuso d'ufficio; nel 2017 7.000; poi 6.000, poi 5.000. Probabilmente, sarebbero diventati 4.000 e poi 3.000, perché questo era l'andamento naturale. Bastava saper numero di procedimenti che rappresentano quanto? Centinaia di migliaia di procedimenti penali pendenti nelle aule dei nostri tribunali, che si innescano ogni anno nelle aule dei tribunali. Con una fame di giustizia civile, di sveltezza nella giustizia civile, con una fame di personale, una fame di informatizzazione, una fame di assunzioni, noi ci concentriamo su quella che arriva oggi in Aula come se fosse una grande riforma.

sia in contrasto con le previsioni dei trattati internazionali e quindi con l'articolo 117 della Costituzione, che prevede che l'Italia si adegui agli obblighi e alle normative europee e internazionali. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione ONU di Merida che disciplina gli strumenti di contrasto alla corruzione. Tra questi, c'è assolutamente un obbligo che va in questa direzione, di non creare disparità di trattamento e di poteri difformi tra un cittadino e l'altro. Specialmente chi esercita cariche pubbliche dovrebbe avere un *surplus* di responsabilità, non un *minus* di responsabilità. Siccome il problema dei sindaci era già stato abbondantemente risolto, non ne voglio nemmeno parlare: appunto perché il problema era già stato abbondantemente risolto. Il problema dei sindaci essenzialmente, come sa chiunque abbia amministrato un qualsiasi Comune, è ormai un problema di responsabilità erariale,

Innanzitutto, come per tutte le leggi, si fanno per attuare i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di certezza dei loro diritti, di protezione dall'abuso di chi ha una posizione di potere dominante. Invece, qui abbiamo una soluzione che va in senso contrario di quello che ci proponiamo con il dettato costituzionale, con criticità sollevate dai magistrati. Quindi, questo provvedimento solo allo stare dentro le mura dell'ospedale psichiatrico, ma anche a continuare a non ascoltare le voci di chi ci dice che

che non è del tutto forte: può arrivare un'influenza e potremmo ammalarci di polmonite, perché non siamo un Paese robusto. Per diventare un Paese robusto dobbiamo fare riforme strutturali riforme strutturali di semplificazione e di velocizzazione dei processi. Quindi, l'azione fondamentale di questo Governo dovrebbe essere quella di continuare a percorrere la strada del PNNR, perché ancora una volta - sempre ricordando l'esempio delle scarpe

solo nell'ultimo anno, del processo penale e la durata media dei processi è scesa al di sotto della soglia dei 1.000 giorni. Risultati analoghi li avevamo osservati subito dopo l'approvazione della riforma del ministro Orlando. Non c'è stata solo la riforma Cartabia, infatti, ma anche il ministro Orlando aveva messo mano al processo civile. È un abbattimento importante. Allora, perché perché ci troviamo oggi a discutere e continuiamo a discutere, quando parliamo di giustizia, di cose inutili? Prendiamo questo maledetto aereo, signor Sottosegretario, signor Vice Ministro,

delle questioni, dimenticando e omettendo il 99 per cento. Con questo provvedimento noi non stiamo facendo quello che dovremmo fare e dovremmo avere l'ambizione di fare, specialmente con un Governo politico. presidente Bongiorno, finalmente, dopo un anno e mezzo di provvedimenti che non ci hanno convinto moltissimo che hanno introdotto 15 nuovi reati, noi di Italia Viva vediamo la luce rispetto a un atteggiamento un po' troppo legato a trovare la soluzione dei problemi, aggiungendo reati e pene, cercando invece ora di ridisegnare il sistema giudiziario. Io sono un avvocato e, quindi, sono oggettivamente di parte e lo dichiaro. Ho sentito colleghi parlare della giustizia giusta. Io non ho le competenze per parlare della giustizia giusta, ma posso parlare solo della giustizia che ho visto, della giustizia che ho frequentato, delle carceri che ho visto quando ero praticante e che mi hanno indotto a lasciare il diritto penale per fare diritto civile e amministrativo, perché per me era troppo forte vedere persone private di libertà, che erano innocenti ed erano in carcere. Non ce la facevo, forse ero troppo giovane, oggi probabilmente cambierei la scelta, ma all'epoca non ce la feci. Posso raccontare cos'è il diritto amministrativo vissuto, o cos'è il diritto civile, e che non si tratta proprio dei numeri detti in quest'Aula, neanche dopo la riforma Cartabia; per esempio che non c'è più un dibattimento nel processo civile, davanti a un giudice, e tutto ormai è *online*, tutto è inviato per scritto e questo fa molto la differenza anche rispetto all'esito del processo. Chi parla di volare in alto, vorrei che lo facesse. Nel 2021 indagati per abuso d'ufficio sono stati 5.418 (mi dispiace dare un dato del 2021, non ce l'ho del 2023): archiviati 4.613;

(27 condanne e 35 patteggiamenti) sono lievi, perché lieve è il reato, né è tale da portare, per fortuna, in carcere. Tutti questi numeri sono persone che per un po' sono state nelle grinfie della giustizia, senza contare il tempo e il denaro, e sono state spesso oggetto di articoli, perché un articolo non si nega mai a nessuno, soprattutto se queste persone erano sindaci. Per caso questo non è un abuso? *(Applausi)*. Ricordo soltanto dei colleghi come Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, che è stato denunciato per abuso d'ufficio da una sigla sindacale che non era stata invitata a un tavolo; o il sindaco Merola, di Bologna, che fu denunciato per abuso d'ufficio per aver trascritto, quando non era ancora legale farlo, i figli di una coppia omogenitoriale. Allora sarà per quello che, a forza di volare in alto, il Partito Democratico si è dimenticato dei suoi amministratori che hanno chiesto tutti in coro di approvare la legge sull'abuso d'ufficio. Vorrà dire che sono tutti responsabili di abuso d'ufficio o che forse sono preoccupati da come l'abuso d'ufficio si configura oggi? Hanno cercato di cambiarlo tutti, dal 1930 ad oggi, e non ci si è riusciti, evidentemente perché l'aleatorietà del reato contestato fa sì che tutti ci possano rientrare, anche chi non ha invitato una sigla sindacale; anche chi ha deciso di fare una trascrizione forse prima del tempo, seguendo la propria coscienza da sindaco. Poi magari, fra cinque anni, proprio per questo atto, non verrà più riconfermato in carica, ma avrà diritto di fare il sindaco, un sindaco?

considerato e si deve comunque trovare una soluzione. Quando si entra nella gogna, soprattutto mediatica, non si riesce più a tornare indietro. Io sfido chiunque in quest'Aula

Etruria. La sua posizione è stata archiviata su tutto. Ma qualcuno si ricorda di quell'archiviazione o si ricorda piuttosto dei giornali che invece lo avevano già condannato? E allora, sì, siamo felici che finalmente sia arrivato un provvedimento che mette un po' di ordine, anche per un tema che a me sta molto a cuore, quello della giustizia preventiva con l'arresto,

è in carcere, in attesa di essere giudicato. Quando si parla della Costituzione del Novecento, nata dopo il buio

ristretta solo in casi eccezionali. E invece in questi anni abbiamo vissuto la restrizione della libertà come mezzo per fare confessare le persone, per fiaccare lo spirito,

per cercare di avere determinate conseguenze. Senza che nessuno si senta escluso perché - come diceva il poeta - la storia dà torto e dà ragione, tutti noi che facciamo politica e abbiamo l'orgoglio e la fierezza di farlo - immagino che nessuno sia qui per caso, ma perché ha una passione e delle idee da manifestare - ci dobbiamo ritenere responsabili di avere per troppo tempo lasciato che la magistratura adempisse

riempire il vuoto quanto basta, perché quanto basta non esiste mai, perché c'è sempre un vuoto da riempire e, quando la politica è debole, lascia che siano altri quei vuoti. Saranno dei titoli di giornale o sarà chi si occupa di quello che dovrebbe essere un potere indipendente rispetto alla politica e che invece per molti anni è stato anche strumentalizzato dalle forze politiche da una parte e dall'altra - quindi tutti siamo responsabili - per fare opposizione? Se veniva inquisito il tuo avversario politico, godevi perché pensavi di poter vincere le elezioni politiche la volta dopo, e anzi utilizzavi quelle indagini

sarà anche interessante fare un'analisi di quella che è stata, da "Mani pulite" in poi, la giustizia, senza essere troppo qualunquisti e gettare la spugna dicendo che è stato

- e dovrebbe farlo - è che utilizzare le indagini per affossare i politici di turno porta male alla politica in genere. Poi c'è il rischio che questa ruota prima o poi giri e tocchi a quello che il giorno prima godeva perché l'avversario politico era finito sotto la gogna mediatica di doversi giustificare in pubblico, nessuno escluso. *(Applausi)*. È per questo che, sebbene ci aspettiamo ancora di più, nel senso che questo è l'inizio di un cambiamento complessivo nelle politiche della giustizia - so che posso parlarne a una persona che la pensa come me

diretta a intervenire in maniera decisiva su quello che è stato ed è uno dei problemi più gravi del nostro Paese: la cronica lentezza dei processi. Una giustizia lenta è sempre una non giustizia, una giustizia denegata. Così ha dichiarato il Ministro nelle sue comunicazioni al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, ricordando l'impatto negativo dei ritardi della giustizia che ci costano due punti di PIL. Ebbene, apprezziamo la consapevolezza mostrata dal Ministro, ma di certo questo disegno di legge non è la soluzione al problema. Si tratta invece di interventi settoriali - chirurgici potremmo dire - attraverso i quali si modifica la disciplina finora vigente in ben tre ambiti diversi. Punto primo: si cancella il reato di abuso di ufficio e si depotenzia fortemente il reato di traffico di influenze illecite. Punto secondo: si interviene pesantemente sulle intercettazioni, limitandole sia nell'utilizzo dello strumento da parte dei pubblici ministeri, sia vietandone la pubblicazione in una serie di casi, con buona pace della libertà di stampa. Punto terzo: si prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento limitatamente ad alcuni reati. Questa previsione - secondo una parte degli auditi - pone persino questioni di compatibilità costituzionale, e lo sappiamo. Voglio soffermarmi ora in particolare sui primi due punti, che ritengo di interesse essenziale per comprendere e criticare il piano del Governo in materia di giustizia. Sull'abuso d'ufficio, nonostante le illustri critiche mosse al provvedimento nell'ambito delle varie audizioni, la Commissione ha ritenuto di non apportare modifiche al testo originale. Il risultato è che, con l'approvazione definitiva del disegno di legge, il reato di abuso di ufficio verrà espunto dal nostro ordinamento penale, unico caso in Europa. La relazione al disegno di legge motiva l'intervento abrogativo con la considerazione che il numero delle condanne dibattimentali per abuso d'ufficio è particolarmente basso, mentre il numero delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato è alto, e queste perlopiù danno luogo ad archiviazioni, come diceva la collega prima di me. Il che comporterebbe, quindi, uno spreco di risorse da un lato e, dall'altro, la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali in particolare. La relazione, però, non considera che la definizione con provvedimento di archiviazione non comporta, di regola, un rilevante dispendio di risorse. Inoltre, ben più importante da considerare è che l'abolizione del reato farebbe venir meno il disvalore sociale che i fatti penalmente illeciti sul piano internazionale hanno per il nostro ordinamento

intenzionalmente siano state economicamente vantaggiose per l'autore o ingiustamente dannose per altri. Qual è il significato del messaggio che diamo alla collettività nazionale e quale l'effetto nei rapporti internazionali, a fronte, tra l'altro, della convenzione ONU contro la corruzione che impegna gli Stati membri a prevedere come reato l'abuso d'ufficio? Non è un caso che una delle prime critiche alla decisione di questo Governo di abrogare il reato di abuso d'ufficio sia arrivata proprio dalla commissaria agli affari interni dell'Unione europea, la svedese Ylva Johansson, che, a settembre dello scorso anno, è tornata ad avvisare il Governo italiano sui rischi che le modifiche normative in questione possano influire sull'efficacia dell'individuazione e del contrasto della corruzione, e ha ribadito, inoltre, che il reato d'abuso d'ufficio è uno strumento importante, anche perché riguarda l'esercizio di funzioni pubbliche per conseguire un vantaggio personale. Come si comprende facilmente, il messaggio che rischiamo di trasmettere ai cittadini è che i loro diritti dipendono dalle intenzioni di chi occupa una posizione di potere. Questa visione trova conferma nel depotenziamento che il cosiddetto disegno di legge Nordio, senza ragione, rivolge anche al delitto di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, ovverosia il traffico di influenze illecite che, introdotto nel 2012 con la riforma Severino, ha poi nel 2019 inglobato il millantato credito, di conseguenza abrogato. Il traffico di influenze illecite conteneva, sino ad oggi, anche una ipotesi di frode rappresentata, appunto, dal previgente millantato credito, per cui la prospettiva di eliminare dal delitto di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale l'ipotesi di frode originariamente classificata come millantato credito non fa altro che depotenziare ulteriormente e in modo del tutto irragionevole (rilevante anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione) la tutela penale della pubblica amministrazione (rilevante anch'essa a livello costituzionale *ex* articolo 97) sotto il doppio profilo dell'imparzialità e del buon andamento, rilevanti sia sotto l'aspetto dell'abuso d'ufficio che su quello del traffico di influenze illecite. In conclusione, in particolare su questo punto, la riforma ha l'obiettivo anche se non dichiarato, di voler sensibilmente indebolire la lotta alla corruzione. E la prova lampante è data dal fatto che è stato bocciato senza appello il nostro emendamento che ha riproposto il testo predisposto dal professor Tullio Padovani nel 1996 per la commissione di studio presieduta presieduta da Giuseppe Morbidelli che, al fine di rendere la fattispecie di reato più definitiva e più tassativa, propone lo spacchettamento dell'abuso d'ufficio in tre distinte ipotesi criminose: prevaricazione, favoritismo affaristico e sfruttamento privato dell'ufficio. Vi avevamo offerto la soluzione al problema, ma non l'avete neanche presa in considerazione, perché la verità è che preferite creare una sacca di impunità. È opportuno, infine, fare un ultimo passaggio sulle intercettazioni. La scelta del Governo di intervenire su due fronti, impedendo - da un lato - al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardano soggetti diversi dalle parti e - dall'altro - vietandone la pubblicazione, indebolisce ulteriormente il ruolo della legge nei confronti di chi riveste riveste incarichi di potere. Anche in questo caso il portato di questa legge e insieme il messaggio che quest'Assemblea, votandola, manda all'opinione pubblica sono molto chiari: è un ostacolo nei confronti della magistratura, un bavaglio nei confronti della stampa, un regalo a chi vuole approfittare della sua posizione pubblica per interessi privati. La verità è che, quando questo disegno di legge diventerà legge, l'Italia sarà un Paese in cui questo abuso sarà non solo consentito, ma legittimato. L'effetto è chiarissimo: un passo indietro nel rispetto dei diritti di chi non ha potere; un passo indietro per tutta la nostra democrazia,

Signor Presidente, approda in Senato un provvedimento che l'Italia e gli italiani aspettavano da tanto tempo, un provvedimento che riporta il cittadino al centro dell'azione politica del Governo. Si dice che la giustizia sia come un treno sempre in ritardo: in ritardo sui processi che dovrebbero marciare spediti; in ritardo nella realizzazione di tutele e garanzie nei confronti dei cittadini; in ritardo nella rimozione degli ostacoli che impediscono sia al mondo giudiziario che a quello amministrativo di essere efficienti e in ritardo, soprattutto, nel riformare la giustizia e renderla davvero giusta ed etica per il cittadino che - ricordiamo - è uguale ad ogni altro davanti alla legge. un provvedimento che ricalca uno dei valori che rappresenta l'identità del Gruppo Forza Italia, il garantismo. È proprio in un'ottica puramente garantista che si incardina questa riforma della giustizia tanto voluta dal presidente Berlusconi e dal senatore Niccolò Ghedini. *(Applausi)*. Oggi siamo qui per approvare un disegno di legge che comincia a restituire al Paese principi di civiltà giuridica, che negli anni erano andati perduti provocando profonde ferite sulla pelle degli italiani. Quello che stiamo facendo è un lavoro complesso per realizzare un preciso impegno che abbiamo preso con i nostri elettori. È un lavoro che il ministro Nordio sta svolgendo con straordinaria tenacia, nonostante chi, in servizio permanente effettivo, continua a screditarlo. Noi siamo a fianco del Ministro e andiamo avanti su questa strada che è tracciata, perché queste battaglie sono le nostre storiche battaglie. Veniamo quindi al disegno di legge. Prima di tutto era doveroso intervenire sulle emergenze; poi, in una successiva fase, riorganizzeremo in modo organico l'intero apparato giudiziario, adeguandolo ai tempi moderni per tenere il passo con le grandi democrazie occidentali e garantire la certezza del diritto, intesa come infallibilità, ma come regolarità e tempestività nelle procedure e nei processi. Le lentezze, le lacune e le inefficienze della macchina giudiziaria costano al nostro Paese, alle imprese italiane e ai cittadini oltre due punti di PIL, cioè più di una manovra finanziaria. Come non definire un'emergenza la doverosa abolizione dell'abuso d'ufficio? Un reato che, nei fatti, ha ingolfato il motore amministrativo del nostro Paese ed è servito soltanto come testa d'ariete per demolire carriere, storie umane e politiche, onorabilità. Gli amministratori venivano intrappolati nelle maglie della giustizia in processi senza fine, per poi venire assolti nella quasi totalità dei casi. Nel 2021, solo per fare un esempio, per l'abuso d'ufficio è stato archiviato l'85 per cento cento se consideriamo assoluzioni e proscioglimenti. In altre parole, era un reato inutile e noi lo abbiamo abolito; era un reato dannoso perché incuteva il timore di agire, la cosiddetta paura di firma, minando inesorabilmente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Non parliamo di una battaglia ideologica del centrodestra, perché i sindaci che hanno fatto la fila per chiederne la cancellazione hanno tutti i colori politici e spesso si sono messi in contrapposizione con i partiti di appartenenza. Noi li abbiamo ascoltati. Noi abbiamo ascoltato il Paese. Urlate che ci mettiamo contro l'Europa, ma urlare non significa dire la verità; anzi, di solito, più si urla e più si mente. Infatti l'Europa non ordina, invita semplicemente a prendere in considerazione. Noi lo abbiamo fatto e siamo venuti alla conclusione che l'abuso d'ufficio ha provocato solo danni. Discorso analogo va fatto per il traffico di influenze, che abbiamo modificato dopo che il ministro Bonafede l'aveva stravolto in senso giustizialista, prevedendo che bastasse anche solo la mediazione per finire sotto inchiesta, portando le lancette della democrazia e dello Stato di diritto indietro nei secoli. A proposito di tentativi di riportare indietro l'orologio all'epoca dei fustigatori, c'è chi delle opposizioni cerca di convincerci che regolamentare la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni, vietare di intercettare le comunicazioni fra un indagato il suo difensore, vietare il sequestro dei telefonini, siano un modo per mettere il bavaglio alla stampa e intralciare le inchieste e il corso della giustizia. Al contrario, sarebbe grave e colpevole non intervenire di fronte a chi trova legittimo intrufolarsi e scandagliare la vita privata delle persone, guardare dal buco della serratura *(Applausi)*, a maggior ragione se estraneo a un'inchiesta e senza proteggere il diritto alla riservatezza nei nei rapporti tra avvocato e cliente. Infatti, con questo provvedimento cambia la prospettiva con cui guardiamo a questo diritto fondamentale e finisce il Bronx delle intercettazioni affidando al solo giudice l'individuazione di quelle pubblicabili. ed elementare, colleghi, ed anche un bambino capirebbe questa logica che ha a che fare con il diritto, con la giustizia, con la libertà di ogni singolo individuo. Fa finta invece di non capire chi ogni giorno grida e invoca quella libertà di stampa che, per fortuna, nel nostro Paese è totale e senza limiti. Andate a fare un giro in altri Paesi a voi così affini, come la Cina *(Applausi)*, per vedere cosa significa censura e bavaglio ai giornalisti. Se la pubblicazione delle intercettazioni a strascico è barbara, il sequestro dei telefonini è una pratica addirittura selvaggia, alla quale giustamente poniamo rimedio. Non possiamo negare che nei nostri cellulari è custodita tutta la nostra vita: non solo le conversazioni private, ma foto, dati sensibili come le cartelle cliniche, risultati di analisi (spesso anche di terze persone). Frugare nella nostra intimità è aberrante e noi a questa aberrazione poniamo la parola "fine". Stiamo lavorando per mettere alle spalle oltre un trentennio nel corso del quale la giustizia è diventata un tritacarne, nel quale un cittadino sa quando ci finisce dentro e ignora quando ne esce, con la sola consapevolezza che potrà rivedere la luce solo dopo tanto, tantissimo tempo; una sorta di fine processo mai. Non a caso, per i reati minori, quelli che prevedono una pena fino a quattro anni, escludiamo la possibilità che, in caso di assoluzione, il pubblico ministero una storica battaglia del presidente Berlusconi che tuttavia riteneva, a ragione, che questa norma di civiltà riguardasse tutti i procedimenti. Ma sono certa che prima o poi ci arriveremo. In tutti questi anni si è cercato di capovolgere l'onere della prova, si è diventati tutti presunti colpevoli. Le norme a garanzia degli imputati sono diventate condanne mediatiche anticipate. Le ordinanze di custodia cautelare sono usate per stravolgere confessioni e spesso sono fondate su elementi inconsistenti. È questo il motivo per cui, quando si vuole spedire in carcerazione preventiva un indagato, introduciamo l'obbligo dell'interrogatorio preventivo, non dopo cinque giorni in cella, ma prima di finirci; e non sarà un giudice solo a decidere, ma sarà un collegio di tre giudici. Onorevoli colleghi, noi sentiamo sulle spalle il dovere, la responsabilità di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e la giustizia. La politica di questo Governo e di questa maggioranza è molto chiara: lo Stato deve essere severo con chi sbaglia, deve punire chi viene condannato da una sentenza definitiva, ma deve anche essere in grado di assicurare il rispetto delle garanzie del giusto processo, altrimenti diventa un aguzzino. un aguzzino. La riforma della giustizia penale, che come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto, in questo provvedimento riesce in un'impresa molto semplice, anche se talvolta è la più difficile da compiere: garantire i diritti del cittadino in virtù dei principi costituzionali. È un primo passo e tanti altri ancora devono essere fatti anche per migliorare questa riforma. Ogni processo che dura troppo tempo e ogni errore giudiziario rappresentano una sconfitta per tutti noi, ma non abbiamo alcuna intenzione di perdere questa battaglia. Stiamo compiendo un'opera grande, che molti credevano impossibile, ossia quella di riformare la giustizia, ma la strada è ancora molto lunga. Abbiamo davanti sfide importanti, una su tutte la separazione delle carriere, che Forza Italia vuole realizzare. Questo è un Governo nato dal consenso popolare e, con la stessa determinazione con cui ha governato finora, riuscirà a tener fede al proprio mandato elettorale, avendo come unica stella polare la difesa e la tutela dei diritti dei cittadini.

intervengo per ultima per il mio Gruppo, come Capogruppo della Commissione giustizia, perché dovrei fare una sintesi degli interventi di tutto il mio Gruppo e dare riscontro a tutti gli interventi che ho Ma non giriamoci attorno: questa riforma per me è veramente un pasticcio. *(Applausi)*. Ho visto la veemenza con la quale ha parlato prima di me la senatrice Ronzulli: il disegno di legge cosiddetto Nordio secondo noi presenta problemi rilevanti (volevo informarla di ciò) e pone quesiti per me allarmanti. Proprio nel momento in cui si dovrebbero restringere le maglie volte al contrasto dei fenomeni corruttivi, in ragione della messa a terra del PNRR, voi abrogate l'abuso d'ufficio, allentate le intercettazioni relativamente alla loro trascrivibilità, depotenziate il traffico di influenze e riproponete, tramite il divieto di appello del pubblico ministero, una sorta di legge Pecorella riveduta, ma non corretta, e comunque forse non sufficiente ai fini del superamento di un eventuale scrutinio di costituzionalità, proprio quando invece servirebbe implementare tutti i meccanismi a protezione dell'ordinamento oramai improcrastinabili, un aggiornamento della disciplina relativa al conflitto di interessi e l'istituzione di un'efficace normativa sulla regolamentazione delle *lobby*. Certo lo impone anche, purtroppo, la cronaca quotidiana. A corollario di ciò - permettetemi giusto una parentesi - sarebbe necessaria anche una riflessione generale sul ruolo da destinare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari anticipato la mia collega Di Girolamo). Siamo proprio sicuri che risponda ancora al suo ruolo di organo paragiurisdizionale, quale giudice terzo ed imparziale nel giudicare i casi che le vengono sottoposti? Siamo sicuri che non appaia invece come un organo politico, oramai desueto, che, in ragione del peso interno dei diversi Gruppi parlamentari, giudica sulla base di valutazioni che a volte esulano dal dato prettamente giuridico? giusto una parentesi, ma ora ritorniamo in merito all'abuso d'ufficio. Questo reato contempla ad oggi una condotta già di per sé molto circostanziata, al punto da confinare la rilevanza penale alle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, cioè i cittadini, lasciati senza protezione nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Pensate soprattutto a loro quando voterete per l'abrogazione, che comporterà l'abolizione di questo perno nella lotta alla corruzione, danneggiando lo Stato e la credibilità delle istituzioni, senza considerare che sul piano strettamente giuridico determinerà effetti pericolosissimi, in quanto ne conseguirebbe l'inevitabile revoca delle sentenze di condanna già pronunciate. Assurdo! Prevedete la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della custodia cautelare in carcere, differendone l'entrata in vigore di due anni, al fine di consentire l'assunzione di 250 magistrati da destinare alle funzioni giudicanti; l'ennesima norma da inserire nel milleproroghe per disporne il ritardo dell'efficacia *sine die*. Inoltre, sapete bene che le incompatibilità derivanti dalla procedura collegiale, estendendosi anche agli altri stati del procedimento, comporteranno quasi una paralisi dell'attività giurisdizionale dei tribunali, a fronte di così poche assunzioni. Abbiamo una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Per questo non abbiamo minimamente compreso la ritrosia nell'approvare il nostro emendamento, che prevedeva l'aumento a 500 magistrati della pianta organica. Senza parole! modo, non abbiamo capito il motivo per il quale non sono stati presi in considerazione emendamenti che prevedevano l'assunzione di personale amministrativo al Ministero e al

Abbiamo un'emergenza in corso, quella delle carceri. Permane, purtroppo, una situazione di sovraffollamento: 51.179 posti disponibili a fronte di 62.707 reclusi, di cui 2.541 donne. Il ministro Nordio, durante l'esposizione delle linee programmatiche relative al Dicastero, ha tranquillizzato sui numeri relativi ai suicidi in carcere. Qui non si tratta di numeri, ma di persone affidate alla custodia dello Stato,

La situazione, nonostante le rassicurazioni del Ministro, riferita anche in occasione del *question time*, dev'essere assolutamente risolta. Anche il Presidente della Repubblica si manifesta preoccupato per la situazione nelle carceri, tanto da sentire il dovere di convocare al Quirinale sul punto il capo del DAP, il pm Giovanni Russo. Tornando a noi, giusto per evidenziare come si è costretti a lavorare in Commissione, lì è stato approvato, con riformulazione, un emendamento volto a rafforzare il divieto di intercettazione, tra l'altro già previsto dall'ordinamento, tra difensore ed indagato. Orbene, il medesimo oggetto vede un disegno di legge in corso d'esame in Commissione, peraltro con emendamenti già presentati e solo da votare. Quando abbiamo riferito dell'inammissibilità o quantomeno dell'inopportunità di tale emendamento, nessuna spiegazione ci è stata data. Tanto, non vi era bisogno di una spiegazione: quello che non può entrare dalla porta, entra da una finestra o, per meglio dire, entra da un'altra porta, giusto? Purtroppo, la china che sta prendendo questo Governo non ci convince, non solo relativamente alla giustizia. State barattando il futuro di questo Paese con la sopravvivenza della vostra coalizione. Potrei dire che stiamo assistendo a una sorta di lottizzazione dei provvedimenti. Autonomia differenziata alla Lega, premierato a Fratelli d'Italia, che anzi, dopo l'approvazione dell'autonomia differenziata, chiamerei fratelli del Nord Italia.

Ne siamo certi: la finta compattezza che state dimostrando con l'approvazione di questi provvedimenti si scioglierà come neve al sole una volta passate le elezioni europee. Allora getterete la maschera e i nodi verranno al pettine. Signor Presidente, spero vivamente che l'approvazione del disegno di legge in esame faccia da spartiacque nell'azione della maggioranza in materia di giustizia. Ripensateci: fermatevi e date retta a quanto scritto nella lettera dei presidenti delle Corti d'appello. Fermatevi sulla prescrizione. Date retta, se non a noi, all'Europa, quando vi chiede di mantenere inalterato l'abuso d'ufficio, così come novellato dal Governo Conte II. Date retta al CSM, quando vi impone di ragionare sulla separazione delle carriere. Altrimenti, darete retta ai cittadini, che a breve inizieranno a chiedere il conto. *(Applausi)*.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

Presidente, onorevoli colleghi, vorrei cominciare questo mio breve intervento ringraziando The Restorers, cioè Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Macrine Atieno e Ivy Akinyi, le cinque studentesse keniote che nel 2019 hanno sviluppato un'applicazione per aiutare le vittime e le potenziali vittime della mutilazione genitale femminile, arrivando nella rosa dei finalisti per il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Le ringrazio qui oggi perché sinora in pochi l'hanno fatto, perché il loro è stato un atto innovativo, a suo modo dirompente e, seppur meritevole, ad oggi poco conosciuto. L'*app* iCut è stata anche un gesto di coraggio e di libertà, considerando la tradizione culturale locale che queste cinque ragazze hanno dovuto sfidare. Nonostante il Kenya infatti le abbia vietate nel 2011,

invita non solo i più giovani, ma anche tutti noi a svolgere un ruolo attivo nella propria comunità contro questo abominio. Secondo gli studi dell'ONU, questa pratica criminale è diffusa ancora in oltre 30 Paesi si stima che quattro milioni di ragazze nel mondo siano minacciate da questa barbara usanza ogni anno e costrette a subirla come un rito di passaggio verso la femminilità matura. La mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani, mette a rischio ogni anno più di 3 milioni di ragazze e bambine: oltre 200 milioni di donne oggi nel mondo vivono le conseguenze di quest'atroce sevizia. Questo implica che entro il 2030 più di una ragazza su tre nascerà in regioni dove questa pratica primitiva è prevalente, con la conseguenza che almeno 68 milioni di ragazze saranno a rischio. pratiche magiche e riti arcaici che si perdono nella notte dei tempi, di cui non è facile ricostruire l'origine, ma delle quali certe sono solo le conseguenze:

un gesto di prepotenza, un'operazione criminale e un atto contro l'integrità del corpo, la dignità della persona e la vibrazione dell'anima, che tutti siamo chiamati a condannare, ancora una volta, fino a quando ce ne sarà bisogno. In occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili voglio perciò riaffermare che l'Italia conferma il suo forte impegno per la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e sulle bambine, come rappresentato anche da una delle priorità del mandato che abbiamo come Paese nel Consiglio dei diritti umani presso le Nazioni Unite. In Italia abbiamo un'ottima legge, la legge Consolo, che è presa ad esempio come *best practice* in altre Nazioni, ma le pene non sono sufficienti. Signor Presidente, bisogna cambiare questa macabra prassi attraverso un incisivo cambiamento culturale nei Paesi d'origine. Dobbiamo condividere il nostro impegno con la società civile e con tutte le istituzioni interessate. Ben vengano perciò progetti educativi, alcuni già in atto in quei Paesi, che promuovano la conoscenza della sacralità del corpo e della donna stessa, affinché alla cultura della violenza si sostituisca quella del rispetto

perché si crei nel lungo termine una coscienza comune più forte della tradizione criminale e cresca una nuova generazione di uomini e donne liberi. Concludo dicendo che non serve essere mutilata per dimostrare di essere una donna.

di una cosa chiamata "detenzione amministrativa", che è un vero e proprio mostro giuridico. Vorrei infatti ricordare che l'articolo 13 della nostra Costituzione dice che la libertà è inviolabile e può essere limitata soltanto con un provvedimento del giudice. Invece noi teniamo

senza che abbiano commesso alcun reato, nell'attesa di essere rimpatriate verso Paesi dove non saranno mai rimpatriate, per il semplice motivo che non abbiamo accordi di rimpatrio verso quei Paesi. Così succede che un ragazzo di ventidue anni che si chiamava Ousmane Sylla - lo voglio ricordare con nome e cognome perché è giusto così e che il suo nome risuoni

la cosa più dignitosa che potremmo fare noi italiani è esaudire il desiderio di questo ragazzo, che si è tolto la vita per essere stato messo in una condizione che un Paese civile non dovrebbe accettare. Questo suicidio si aggiunge ai 15 che abbiamo avuto nei nostri penitenziari, cinque soltanto nella casa circondariale di Verona in un anno, praticamente una strage. Continuiamo ad avere una lunga scia di sangue anche perché, come nei CPR, anche nelle nostre carceri le condizioni di vita non sono dignitose. Dire che costruiremo nuove carceri non risolve il problema. Vado a chiudere perché, al contrario della collega di Fratelli d'Italia, rispetto il tempo. Dire che costruiremo nuove carceri non è una risposta, perché le nuove carceri saranno pronte, se va bene, tra dieci anni. Nel frattempo, abbiamo un numero di

rendere un'informativa per spiegarci cosa intende fare per evitare che il nostro Paese subisca ancora l'onta di una condanna a livello internazionale perché purtroppo riserviamo più spazio ai suini negli allevamenti, con tutto il rispetto, che ai nostri detenuti nelle carceri patrie.